«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi

senatori, mercoledì scorso si è spento Paolo Rossi, calciatore e opinionista sportivo, ma soprattutto uno dei simboli più emozionanti dello sport italiano. Ricordarne la figura nella solennità dell'Aula del Senato significa per tutti tornare indietro con la memoria a quasi quarant'anni fa, all'immagine di quel ragazzo pulito, garbato, educato che, con incredibile tenacia, coraggio e determinazione, ha infiammato il cuore di un'intera Nazione. Era l'estate del 1982 e i milioni di italiani che hanno invaso le strade e le piazze di ogni dove per festeggiare la vittoria dei Mondiali di calcio in Spagna sono il più bel ritratto di un popolo che nello sport aveva ritrovato tutta la sua forza, tutto il suo carattere e la sua unità. Sono il ritratto di un Paese che, dopo anni di terrore, di sacrifici economici, di scontri sociali e forti tensioni politiche, aveva afferrato un'occasione di riscatto, si riempiva di orgoglio e si candidava a diventare protagonista dello scenario internazionale. E ci riuscì proprio grazie alle prodezze del calciatore italiano con il nome più italiano di sempre, di quel Paolo Rossi che, partendo da una piccola squadra di provincia, un passo alla volta, senza arrendersi mai di fronte a mille difficoltà, ha raggiunto la vetta del mondo ed è diventato un modello positivo dentro e fuori dei campi di calcio per intere generazioni. L'esempio di un Italia concreta, intelligente, creativa, instancabile e generosa. Un atleta che ha fatto sognare l'Italia e che questa Italia non smetterà mai di amare. Per questo è ancora più odioso aver appreso che, proprio durante i funerali, la sua casa di Bucine è stata svaligiata da persone senza scrupoli e senza umanità. Alla moglie Federica, ai figli e a tutta la famiglia desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza del Senato. In ricordo di Paolo Rossi, campione italiano nel mondo di sport e sportività, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Paolo Rossi non è stato solo un grandissimo calciatore e neppure solo un grandissimo sportivo.

e tutti lo ricordiamo nella mitica nazionale del 1982, quella che sabato lo accompagnava in spalla nel suo ultimo viaggio: i suoi fratelli, perché non erano solo amici quelli che avevano condiviso il mondiale più bello che ha unito tante generazioni, ma erano come fratelli. Ricordiamo i suoi gol nella Nazionale, nella Juve, i periodi anche un po' più negativi che ha vissuto nel Perugia e nel Milan. Ma era Paolo Rossi soprattutto nel suo amatissimo Lanerossi Vicenza. Quella Vicenza che lo ha adottato e che gli ha consegnato la cittadinanza onoraria. Quella Vicenza che venerdì, con grandissima compostezza e anche con discrezione - che era poi una delle doti di Paolo - lo ha salutato prima allo stadio e poi durante il suo funerale.

Con chiunque lo avvicinasse era sempre lui, semplice, con il suo sorriso, le sue battute, la sua gentilezza, la sua generosità, quell'altruismo che metteva in campo, nello sport, ma che faceva parte della sua vita. Ha fatto tanto bene, ha fatto tanta beneficenza. Era una persona che credeva molto nella solidarietà e per questo era amato da tutti. Era amato anche da chi non seguiva il calcio. Ognuno di noi, penso di poterlo dire anche a nome di quest'Assemblea, di tutte le colleghe e i colleghi, ha grazie a lui dei ricordi indimenticabili legati alla nostra vita, ad un pezzo di storia di questo Paese. Paolo Rossi era un campione di valori, un fuoriclasse dentro e fuori dal campo. Ci ha insegnato a coltivare il sacrificio e ha sofferto tanto. Ha fatto riscoprire all'Italia di essere una Nazione unita, un popolo che nelle sue emozioni trovava l'identità e la forza di guardarsi e andare avanti, dice il mio amico Fabio Poli dell'Associazione calciatori italiani. Ieri, poi, scriveva questa bellissima lettera aperta il presidente Gabriele Gravina: «Paolo lo ricorderemo per sempre con le braccia al cielo, il sorriso sulle labbra e il Tricolore sul cuore». O ancora, un amico giornalista vicentino, Antonio Di Lorenzo, detto: «non è solo Vicenza che sfila sul verde dello stadio Menti, ma tutta l'Italia». Antonio Cabrini ha detto che Paolo era veloce e se n'è andato così, velocemente, in silenzio. Ma il suo ricordo non morirà mai e non è retorica, perché ha davvero abbracciato tante generazioni Ora, però, sta a noi ricordarlo come avrebbe voluto. Ci saranno molti momenti in cui lo ricorderemo, faremo iniziative e manifestazioni, gli dedicheremo insieme, anche nella nostra città di Vicenza, un luogo importante come lui merita. Le ultime parole le voglio esprimere ricordando e abbracciando anche dall'Aula del Senato la sua meravigliosa famiglia, la splendida moglie Federica, le figlie Maria Vittoria e Sofia Elena e il figlio Alessandro. signor Presidente, dicendo questo: Paolo diceva che la morte è semplicemente spostarsi nella stanza accanto. Ecco, io voglio pensare questo, che Paolo sarà sempre accanto alla sua famiglia e a tutti noi che gli abbiamo voluto bene. Grazie Paolo, ciao Pablito.

ho letto la notizia dell'improvvisa scomparsa del grande calciatore Paolo Rossi, il mio sentimento è stato di incredulità, subito ho pensato a una *fake news* di cattivo gusto, legata alla scomparsa di Maradona. Questo Questo sentimento si è trasformato in un velo di tristezza che mi ha accompagnato per un paio di giorni, quando purtroppo le agenzie hanno confermato la triste notizia. La figura di Paolo Rossi fu indissolubilmente legata al trionfo azzurro del mondiale di calcio di Spagna del 1982, un evento che non fu solamente - l'ha già ricordato il Presidente una grande vittoria sportiva, come ebbe a comunicarci lo storico triplice annuncio di Nando Martellini che eravamo campioni del mondo, ma quella vittoria fu l'emblema di quegli anni Ottanta che chiudevano il periodo più buio del terrorismo e determinarono il rilancio morale ed economico del nostro Paese. Paolo Rossi - Pablito, come è stato ribattezzato - è stato quindi uno dei protagonisti di una tappa significativa della storia italiana del secondo dopoguerra. Egli fu indubbiamente uno dei giocatori più forti in assoluto del calcio mondiale, come fu suggellato dal «Pallone d'oro» del 1982, dai successi nei *club* del Lanerossi Vicenza, Perugia e soprattutto della Juventus. Interpretava il ruolo di attaccante in modo intelligente e astuto. Certo, Paolo Rossi non era il classico centravanti da sfondamento come lo furono Giorgio Chinaglia o Christian Vieri, ma le sue caratteristiche erano la rapidità, il fiuto della posizione giusta al momento giusto, l'agilità, quasi segnasse i *goal* in modo garbato, un garbo che egli ha anche avuto nel lasciare questo mondo, in punta di piedi, con la riservatezza e l'intelligenza che lo hanno sempre contraddistinto, ma davvero troppo presto. Anche il nostro Gruppo porge le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Con te se ne va un pezzo di storia del nostro Paese ed anche una parte importante degli anni spensierati della nostra gioventù. Grazie Paolo, grazie campione del mondo.

Paolo Rossi e, forse, a tutti sarà venuto in mente che in questi anni non abbiamo riconosciuto la grandezza e il valore, non solo sportivo, che che egli ha rappresentato per la nostra Nazione. Fu sicuramente un grande calciatore e, come è stato appena ricordato, fu anche «Pallone d'oro», capocannoniere ai mondiali del 1982, vinti dall'Italia,

andò oltre l'aspetto sportivo. Nel 1982 l'Italia era ancora con i postumi, forse neanche con i postumi, ma con la coda del terrorismo nazionale, quello delle Brigate rosse, ed era ancora dietro alle stragi che si erano verificate da non molti anni. Era un'Italia divisa e divisiva in cui - voglio ricordare il Tricolore era visto con diffidenza; chi ce l'aveva, lo teneva nel cassetto. Chi ce l'aveva, a volte era guardato con sospetto. Non voglio dire altro per non fare politica di parte in questa occasione.

nel 1982, era bello vedere risvegliarsi attorno al nome di Paolo Rossi un sentimento che accomunava gente di orientamenti politici completamente diversi, tutti col Tricolore in mano. Fu un miracolo. Si parla tanto, giustamente, di quale significato abbia avuto nell'immediato dopoguerra la vittoria di Bartali al Tour de France. Si dice che salvò l'Italia dalla rivoluzione. Io credo che Paolo Rossi fece qualcosa di diverso, ma forse, in un certo senso, più grande perché restituì all'Italia un'anima nazionale. Perché non dire come stavano veramente

Ricordo che quell'estate mi recai all'estero e le persone più umili appena ci vedevano e capivano che eravamo italiani ci urlavano «PaoloRossi», tutto attaccato. «PaoloRossi», tutto attaccato. Era diventato l'italiano più famoso nel mondo e l'italiano di cui essere più orgogliosi nel mondo. Rendo allora a lui un grande omaggio e un grande affetto. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo. Non mi posso definire amico perché l'avrò visto in vita mia al massimo sette volte, ma ho avuto la possibilità di apprezzare il suo modo di essere, la sua semplicità, la sua umanità il suo essere capace di volare alto sulle divisioni. Scusate allora se finisco non con una polemica, ma con un'annotazione necessaria da parte mia e del mio movimento politico. Come avete visto in nessuna dichiarazione abbiamo cercato di mettergli la maglietta politica; eppure lui nel 1999 si era candidato alle europee con Alleanza Nazionale e mai ha rinnegato quella scelta. Mi aspettavo che qualche giornale lo potesse ricordare, cosa che sarebbe successa se si fosse candidato a sinistra. Non ci siamo però lamentati. Mi lamento di una cosa diversa, signor che la Rai, servizio di Stato, in un'edizione straordinaria di «90° minuto» ha ritenuto di invitare, per commemorarlo, Di Maio e uno dei giornalisti non voglio dire più odiosi, dirò qui più divisivi che esistano, come Scanzi, che nulla hanno a che fare - né l'uno, né l'altro - con lo sport e men che meno con Paolo Rossi. Lasciate che Paolo Rossi, come abbiamo fatto noi, che semmai ne avevamo i titoli, appartenga a tutti. Non tiriamo la maglietta a Paolo Rossi, che di maglietta ne ha una sola: quella azzurra con il tricolore stampato sul petto.

in questo drammatico 2020. Lo vogliamo giustamente ricordare in modo così solenne nell'Aula del Senato della Repubblica, perché quest'uomo l'eterno ragazzo con la maglia numero 20 dell'Italia - ha lasciato un segno nella storia recente del nostro Paese. Sì, Paolo Rossi è stato il simbolo di quell'Italia che vinse i Mondiali di calcio del 1982, un campione gentile che con i suoi goal unì un Paese intero e rese felici tutti: amanti del calcio, dello sport e non solo. Fu proprio così, perché rese quell'estate indimenticabile e non è un caso che la sua morte abbia colpito tutti, anche chi nel 1982 non era ancora nato. Che amara coincidenza: se ne sono andati via, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Emanuela Audisio, sulle pagine del quotidiano «la Repubblica», scrive che Paolo Rossi è stato il nostro Maradona, ma alla maniera di Paolo Rossi: due personalità completamente diverse, due calciatori tecnicamente diversi, ma che hanno entrambi fatto la storia recente del calcio nel nostro Paese. Pablito con la maglia azzurra dell'Italia, Maradona con quella del Napoli; Paolo Rossi fermo per due stagioni per lo scandalo del calcioscommesse, Diego Armando Maradona con la sua vita tribolata dagli eccessi. 1982: voglio ricordare quell'estate di trentotto anni fa, perché grazie all'Italia del calcio tornammo a manifestare nelle piazze dietro il tricolore, uniti. Avevamo alle spalle anni terribili e altri ne avremmo vissuti in seguito. Due anni prima c'era stata la strage alla stazione di Bologna, quattro anni prima il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e - ancora - noi napoletani eravamo nel pieno dell'emergenza post-terremoto del 23 novembre 1980. Ebbene, in quell'estate di trentotto anni fa riscoprimmo la felicità e fu proprio il presidente della Repubblica Sandro Pertini a interpretare quel nostro stato d'animo. Quella sua gioia irrefrenabile accanto al re Juan Carlos, al quale disse: «Con questi azzurri non ce n'è per nessuno», lo rese portavoce del nostro sentire comune. Ma come, con tutti i problemi che abbiamo si pensa alla vittoria dei Mondiali di calcio? Questo chiese l'inviato del TG2 Italo Moretti al presidente Pertini, mentre l'aereo presidenziale riportava a casa gli eroi azzurri. Egli rispose: la settimana è fatta di sette giorni e la domenica è fatta per riposare e gioire. Ecco, oggi è domenica, domani sarà lunedì. Presidente, colleghe e colleghi, quella dell'82 non è stata solo la nazionale di Paolo Rossi. Li ricordiamo tutti: Bearzot, Zoff, Tardelli, Bergomi, Cabrini, Graziani, Antognoni, Gentile, Collovati, Scirea, Oriali, Conti. Insomma, vinse un'intera squadra e i componenti di quella squadra sono rimasti amici per sempre e tutti loro, gli straordinari ragazzi dell'82, fanno parte delle nostre vite. Grazie campioni, grazie Paolo Rossi. Signor Presidente, ringrazio la Presidenza per questo momento solenne. C'è un'epica nella vita, e in special modo nello sport, a cui alcuni sono destinati. Paolo Rossi lo è stato. È stato ed è un eroe nazionale, con la naturalezza, con la semplicità, con il sorriso di un ragazzo come un milione di altri, come siamo stati ragazzi noi che andavamo a scuola mezz'ora prima che suonasse la campanella per giocare a pallone nel pezzo di asfalto davanti al portone d'ingresso, con un pallone improvvisato e due pietre o due giubbini messi a terra per segnare i pali della porta; come un milione di noi per tutte le domeniche mattina o i sabati pomeriggio passati su campetti umidi, pieni di fango, che erano la nostra felicità e che sono la felicità dei nostri figli. all'emozione delle trasferte o delle partite in casa, dei campionati dei giovanissimi, degli allievi, della seconda categoria dei nostri paesi, delle nostre

Paolo Rossi fu leggenda molto prima di quel 5 luglio 1982 allo stadio Sarriá di Barcellona, molto prima del mondiale. Diventò leggenda con la maglia della squadra Lanerossi Vicenza, che condusse a pochi minuti dallo scudetto, quando già da ala destra era diventato formidabile e geniale centrattacco e costruttore di gioco, costruttore di spazi, di geometrie in campo come seppe dimostrare ai Mondiali del 1978 in Argentina, dove la maglia azzurra e Paolo Rossi divennero una cosa sola per sempre. Come tutti gli eroi, signor Presidente, cadde e seppe rialzarsi dopo gli infortuni al ginocchio, dopo la gogna ignobile e ingiusta, che non volle mai accettare, dell'inchiesta del calcioscommesse. Fu Bearzot ad aspettarlo e a volerlo ai mondiali di Spagna e arrivò quel 5 luglio

grande quanto un Paese, l'Italia, che usciva da anni bui e tremendi. Quella sera e le successive, è stata carica di gioia e piena di speranza per il futuro, e poté festeggiare con Rossi, con Bearzot con il Presidente Pertini, con tutti i ragazzi del *mundial,* che dovremmo ricordare ad uno ad uno e che qualche giorno fa hanno portato Paolo Rossi a spalla tributandogli l'ultimo commiato. Presidente, ogni storia di calcio è una storia di memoria collettiva, piena di mille altre storie; le storie di ognuno di noi, di un Paese intero, della nostra Italia. Paolo Rossi è il giocatore che ha saputo entrare nella leggenda, il cui nome è impresso nella storia del calcio mondiale e nella storia collettiva di un Paese il nostro -, nella storia familiare e sentimentale di ognuno di noi, di ogni italiano. Osvaldo Soriano, un grande scrittore e un calciatore mancato, ha scritto: ogni volta che entravo in area di rigore avevo l'impressione di guadagnarmi

Il suo sorriso, la maglia azzurra numero 20, le braccia alzate al cielo: è questa l'immagine che rimarrà per sempre con noi. Un grido di gioia: una, due, tre volte, tutte nella stessa partita contro il Brasile; poi, di nuovo, in finale, nella notte magica di Madrid, per trasformare la speranza in un sogno, l'attesa in un attimo unico e irripetibile. "PaoloRossi", tutto attaccato, come lo chiamavano i suoi tifosi, e soprattutto come lo chiamavano sottovoce gli avversari, che lo temevano come nessun altro. Un fisico gracile sin da piccolo, quando sognava di fare l'astronauta, non il calciatore, non un fenomeno di atletica, ma capace di una volontà e di una rapidità straordinaria che gli consentiva di anticipare le mosse degli altri. Il destino nel nome, un nome comune da "signor Rossi", appunto, diventato unico, orgoglio di un Paese e di una generazione. Il Paolo nazionale, il "Pablito mundial", che ci portò in pochi giorni dove nessuno avrebbe nemmeno osato immaginare, perché davanti c'erano i fenomeni, i predestinati: da una parte, avversari che sembravano imbattibili, dall'altra, i nostri ragazzi di Spagna 1982, con quel centravanti apparentemente fragile, in disparte, intimidito da una lunga squalifica, ma pronto a guidare quella che si sarebbe rivelata una riscossa collettiva. La riscossa di un Paese che usciva da lotte sociali, crisi economica, divisioni politiche, dall'insensata temperie del terrorismo. Dai suoi gol, dagli abbracci degli azzurri, dalle bandiere tricolore, dalle feste di piazza l'Italia ritrovò fiducia, ottimismo, la voglia di rialzare la testa e vincere tante sfide, conoscendo un momento di autentica, insperata e totale felicità. Quel momento indimenticabile che tutti noi ricordiamo; ricordiamo dove eravamo, ricordiamo vicino a chi eravamo, come ricordiamo la filastrocca della formazione: «Zoff, Gentile, Cabrini Le immagini di Spagna '82, senza nulla togliere agli altri nostri trionfi sportivi, restano quelle più familiari, perché accompagnate da quel sorriso semplice, fresco, che diceva tutto e univa il Paese, oltre le appartenenze, le rivalità, il tifo, le simpatie. Una prova corale di un gruppo così determinato e affiatato al punto di fare della maglia azzurra l'abito della festa di un Paese intero, che aveva voglia di uscire a gridare la gioia di una comunità ritrovata. Un regalo straordinario in quelle serate di giugno e luglio, un'epifania fuori stagione, il trionfo di un'Italia che si immedesimava in quella Nazionale e nell'esultanza senza freni del suo presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Di quei sentimenti Paolo Rossi è stato l'artefice, come gli hanno riconosciuto gli stessi compagni, inseparabili in campo e nell'amicizia. Da quello spirito di squadra Paolo Rossi ha saputo tirar fuori le energie giuste, anche nei momenti di solitudine, quando sembravano venir meno certezze e solidarietà. Paolo, come amava ripetere nelle interviste, e come ha scritto nel libro sulla sua vita, si rivedeva spesso appoggiato ai bordi del Bernabeu, contento di vedere tutta quella gente felice e spensierata. Ha detto di aver voluto fortemente che quell'attimo non finisse più, che durasse per sempre; ma poi ha saputo risvegliarsi, spogliarsi del vestito del supereroe e tornare a essere un uomo normale, un padre, un marito, ritrovando la felicità e l'attaccamento alla vita, giorno dopo giorno, fino all'ultimo, anche nella malattia. Dal campione all'uomo, la stessa persona ispirata ai valori in cui Paolo ha sempre creduto, a cominciare dalla sua fede, mai esibita, coltivata nella sfera intima, lontano dai riflettori. Un fuoriclasse, mai un personaggio, come ha detto sabato mattina, durante i funerali, don Pierangelo; un uomo sensibile, un campione che si era rialzato dalle cadute e dagli infortuni e che ci ha dato una lezione di forza, dignità e amore anche negli ultimi giorni. Li abbiamo visti i nostri eroi dell'82, ognuno al suo posto, emozionarsi sabato mattina come in campo, con la commozione, lo spirito, la medesima voglia di essere una famiglia. A nome del Gruppo Forza Italia mi unisco con affetto al dolore dei familiari e degli amici tutti, con la commossa partecipazione del nostro Paese, che ha salutato un uomo vero, una persona aperta, leale, ironica, attaccata alle radici della sua Prato, ma capace di farsi figlio anche di altre città: Perugia, Torino, Milano, Verona e la sua patria sportiva, Vicenza. Alla moglie Federica, alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, ad Alessandro e alla mamma Simonetta, il nostro più vivo ringraziamento per aver testimoniato uno stile, una vicinanza, un'unione che dovrebbero esserci di incoraggiamento, anche e soprattutto nella grande prova che stiamo affrontando come Paese, istituzioni e comunità civile, e che dovremo sostenere anche nelle settimane difficili che abbiamo davanti. Ricordandolo in quest'Aula di Palazzo Madama - credo di interpretare il sentimento generale - siamo certi di aver avuto in Paolo Rossi un campione di generosità autentica, coltivata nei valori che contano, che sono e devono essere il vanto della nostra Italia di ieri, di oggi e di domani. Paolo Rossi: una bandiera del nostro essere italiani.

Fin da giovanissimo rivelò un grande talento e giunse a Vicenza che sembrava un ragazzo per giocare nella squadra locale. Ammaliò e conquistò la nostra città con il suo sorriso e la sua semplicità. Paolo Rossi era un ragazzo normale, anche se di straordinario aveva tutto. Era il ragazzo che apparentemente tutti potevano essere: sorridente, fiducioso, generoso, serio negli allenamenti, umile anche di fronte ai grandi risultati, come ha dimostrato nel corso della sua brillante carriera e lontanissimo dai divismi che hanno trascinato molti sportivi. Vicenza ha sempre amato quel ragazzo, poi diventato campione e lui ha sempre amato Vicenza e qui ha tenuto contatti, amici e interessi, tanto da sceglierla come luogo dove celebrare l'ultimo solenne saluto. L'Italia di quei tempi stava cercando di lasciare alle spalle i periodi tormentati degli anni di piombo. Tutto stava rinascendo e, parimenti alla squadra del Vicenza, gol dopo gol, quel mondo ebbe un'accelerazione e tutto divenne possibile. Grazie a Paolo Rossi, il Lanerossi Vicenza salì dalla serie B alla A e poi, in un anno, fino al secondo posto, dietro la Juventus. Fu uno sbalorditivo riscatto calcistico che andò di pari passo con una provincia che in pochi anni si era imposta come capitale dell'oro.

portò al mitico trionfo del 1982 quella squadra cui forse solo noi italiani credevamo. Nella nostra storia quella vittoria fu la prima a essere condivisa da tutti. Erano i bei momenti di quell'Italia; quella che sapeva veramente credere e sperare. Le partite del mondiale erano un modo per stare insieme, tutti trascinati dal grande entusiasmo dei gol di Paolo Rossi e da una forte sensazione di appartenenza alla nostra Nazione. Pablito è stato un grande campione, un grande sportivo appassionato e semplice, di grande dignità e capace. Lui resterà per sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori di italiani. A Vicenza abbiamo pianto tutti la sua scomparsa. Commuovono le immagini delle lunghe file per la camera ardente allo stadio Menti e il cordoglio al duomo di tutta la popolazione. Abbiamo visto i vecchi compagni della grande squadra del 1982 e i grandi amici di sempre portare a spalle il feretro. Non lo scorderemo mai. Lo sport, i giovani e tutti noi abbiamo bisogno di buoni eroi e lui lo era. Buon viaggio, Paolo! Grazie Signor Presidente, membri del Governo, senatrici e senatori, ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduto, a eccezione del senatore La Russa. Avrei tanti elementi per replicare al suo intervento, ma mi astengo per il rispetto del momento.

La rete non offriva ancora tutto ciò che oggi è disponibile e il calcio era l'aggregatore principale che permetteva di discutere in leggerezza. Eravamo tutti allenatori, ognuno con la propria soluzione. Quando giocava la nazionale, però, ci si sentiva tutti dalla stessa parte e le partite erano l'occasione per ritrovarsi. Ricordo benissimo il Mondiale del 1982: le prime tre partite, sotto le aspettative di quell'Italia di Bearzot, non avevano soddisfatto l'opinione pubblica e alcune critiche tiravano per la giacchetta il commissario tecnico perché sostituisse Paolo Rossi in vista delle partite con Brasile e Argentina. Io stesso dissi ai miei amici che se avessimo passato di turno sarei andato di corsa da Sassuolo a Magreta (circa sette chilometri) e ricordo che, quando accadde che superammo il turno, un codazzo di macchine e moto mi seguì nell'onorare l'impegno. Oggi, nel rendere omaggio a un formidabile campione mi chiedo: cos'è il calcio per gli italiani? Competizione, rabbia, rancori, voglia di sfida, grandi gioie, delusioni, tifo sfrenato e tanta, tanta passione. Ci sono moltissimi uomini che hanno alimentato la nostra passione per il calcio, ma veramente pochi sono quelli che hanno unito tutti gli italiani, storicamente divisi tra le loro fedi calcistiche. Paolo Rossi è stato questo: un atleta che ha saputo con le sue gesta trasformarsi nel collante per tutta la società italiana. Del resto, la nostra Nazionale da sempre ha rappresentato il il desiderio di vittoria attorno al quale tutti ci stringiamo indistintamente. Quella dell'Italia è una delle fedi che ci accomuna tutti. Troppo spesso non manifestiamo a dovere la nostra italianità ed è per questo che esistono i Paolo Rossi; i grandi giocatori che ci ricordano quanto amiamo il nostro Paese. Colleghi, fa male ricordare persone che hanno rappresentato tanto nella nostra vita, anche se solo attraverso uno schermo della TV o dagli spalti di uno stadio. Ci sono uomini che hanno arricchito la nostra anima e quando se ne vanno un pezzetto di questa viene strappata via e fa male. Nella vita di Paolo Rossi possiamo leggere tante metafore, tutte inserite all'interno di un'esistenza piena di un grande uomo. Paolo Rossi è stato un uomo che ha saputo rialzarsi più volte. Il suo trionfale Mondiale del 1982 non può e non deve essere letto solamente dal punto di vista sportivo, pur ovviamente eccezionale, ma la sua esperienza umana deve far pensare a quanti durante la loro vita hanno subito delle brusche pause, non sempre dovute alla propria volontà. Lo *stop* di due anni a cui dovette far fronte Paolo Rossi fu per lui un momento molto difficile, ma da uomo forte qual è sempre stato ha saputo ripartire subito, anche con un gol, al suo rientro nelle ultime giornate del campionato del solo il preludio al ruolo da protagonista nei sogni italiani del mondiale spagnolo. Le metafore in Paolo Rossi non finiscono qui: lui stesso nella sua autobiografia si descrive come un uomo normale; non un fuoriclasse, non un atleta dalla prestanza fisica strabordante, ma uno che ha saputo farcela con l'impegno quotidiano e con la forza di volontà: uno di noi insomma. Allora voglio rivolgermi non solo a voi colleghi, ma a tutti gli italiani che oggi stanno faticando in questa crisi: siamo tutti uomini normali, rimbocchiamoci le mani e insieme ce la faremo, come ce la fece Paolo Rossi. Voglio concludere il mio ricordo con una frase dello stesso Paolo Rossi che credo sia più attuale che mai e che deve fungere da monito e da stimolo per tutti noi in questa difficile fase di crisi per il Paese: «si può essere stritolati da qualcosa che ci cattura senza che noi abbiamo fatto nulla perché accadesse. Si può diventare vittime e non riuscire a dimostrarlo». Colleghi, oggi siamo tutti noi vittime incolpevoli di questo virus venuto da lontano. Rialziamoci tutti insieme; magari il 2021 sarà anche di aiuto, con quelle che auspichiamo saranno le "notti magiche" dell'Europeo di calcio in ricordo di Paolo Rossi. Ciao Paolo.

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente

la riunione di un Gruppo parlamentare, le Commissioni non potranno riunirsi dalle ore 9 alle ore 11. Mercoledì 16, alle ore 9,30, saranno discusse mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Dalle ore 15 alle ore 16,30 saranno discussi il rendiconto e il bilancio interno del Senato. L'ordine del giorno seduta di giovedì 17 prevede la deliberazione di questioni pregiudiziali, *ex* articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge immigrazione e protezione internazionale e, a seguire, la discussione del medesimo decreto fino alle ore 20,30, che proseguirà, ove necessario, anche nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dicembre.

n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

carattere progressivo, azioni di sostegno ai settori economici più colpiti dalle restrizioni conseguenti alla pandemia. Si tratta di provvedimenti che hanno seguito l'evoluzione delle difficoltà economiche, approntando risposte in grado di adattarsi alle varie esigenze.

Tali provvedimenti, per le caratteristiche che ho appena riportato, devono essere considerati in maniera organica, ricordando anche che ad essi seguirà a breve un altro decreto-legge, una sorta di ristori il quale servirà a dare un'ulteriore risposta di sostegno al nostro sistema economico e produttivo, con l'obiettivo di sostenere tutte quelle attività che, pur non avendo chiuso, hanno però registrato cali di fatturato, perché fanno parte delle filiere collegate ad attività chiuse. Oggi siamo chiamati in quest'Aula a discutere e votare il disegno di legge di conversione del decreto-legge ristori, che conta su una dote complessiva superiore ai 19 miliardi di euro per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico produttivo. Durante il mio intervento vi illustrerò le caratteristiche della parte del disegno di legge collegata al ristori uno e *bis*. L'altro relatore si occuperà di illustrarvi i decreti ristori-*ter* e *quater*. Con il decreto-legge ristori, il Governo ha inteso potenziare la rete di protezione intorno alle categorie economiche più colpite dalle restrizioni introdotte dal

bisogno di compilare moduli e con incrementi che, rispetto al precedente ristoro del decreto-legge rilancio, arrivano fino al 400 per cento. Le attività commerciali sono state sostenute anche con il riconoscimento di un credito di imposta sugli affitti degli immobili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e con la cancellazione della seconda rata IMU. Sono state sospese le procedure esecutive immobiliari per la prima casa fino al 31 Sono stati previsti aiuti al turismo e alla cultura e stanziate risorse per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Per quanto riguarda il lavoro, è stata prorogata la cassa integrazione per altre sei settimane (fino al 31 gennaio 2021) o, in alternativa, sono state concesse ulteriori quattro settimane di esonero contributivo, prevedendo anche il blocco dei licenziamenti la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori delle aziende interessate dal DPCM per il mese di novembre. Per i lavoratori stagionali, inclusi quelli del turismo, dello spettacolo, quelli intermittenti, i porta a porta e i prestatori d'opera, è stata prevista un'indennità *una tantum* da mille euro. Per chi invece ha usufruito del reddito di emergenza sono state previste altre due mensilità. Per quanto riguarda invece la salute, è stata potenziata la capacità di diagnosi rapida dei casi di positività al Covid-19 tramite lo stanziamento di risorse di un piano per i tamponi rapidi antigenici e sono state previste risorse per permettere a medici di famiglia e pediatri di effettuare tamponi rapidi per velocizzare il tracciamento. Per garantire anche agli studenti meno abbienti di usufruire di PC, *tablet* e connessione alla rete, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni per la didattica a distanza. Per quanto riguarda la sicurezza, sono previste risorse per le Forze di polizia e i Vigili del fuoco e interventi nell'ambito della giustizia, per ampliare e semplificare i collegamenti per i procedimenti penali e civili e per favorire le udienze a porte chiuse nei procedimenti civili e penali. Altri interventi sono previsti sull'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo di contenere i contagi all'interno delle carceri.

con il quale l'Italia è stata divisa in tre zone di rischio legate al Covid-19 e classificate come gialle, arancioni e rosse, decretando la chiusura totale di molte attività in quelle rosse e arancioni. quelle rosse e arancioni. Sono stati previsti contributi a fondo perduto alle attività chiuse in conseguenza di questo DPCM e, allo stesso tempo, sono state potenziate le percentuali di ristoro previste dal decreto ristori. Inoltre, il provvedimento incrementa il numero delle attività economiche identificate attraverso i codici Ateco coperte da contributi a fondo perduto, sulla base del decreto ristori. Per quanto riguarda le imprese e l'economia, in particolare sono previsti per le zone rosse indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti su conto corrente fino al 200 per cento di quanto già erogato per le zone arancioni, una maggiorazione del 50 per cento per gelaterie, bar, pasticcerie e alberghi, che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori, arrivando al 200 Sono inoltre previste proroghe relative agli adempimenti fiscali delle imprese, la cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori delle attività interessate dal DPCM e ricadenti nelle zone rosse e il riconoscimento di un credito d'imposta cedibile al 60 per cento per gli affitti delle attività commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per quanto riguarda il lavoro, sono stati sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive. È prevista l'estensione della cassa integrazione agli assunti dopo il 13 luglio 2020. Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, invece, è stato previsto il congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole per i genitori degli alunni delle secondarie di primo grado e il riconoscimento del *bonus* *baby-sitting* per le famiglie residenti nelle Regioni in zona rossa. È stato inoltre istituito il fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e sono state stanziate risorse per il finanziamento dei CAF coinvolti nella lavorazione delle dichiarazioni indispensabili alla fruizione delle varie prestazioni sociali agevolate. Per il potenziamento a incremento del fondo creato dal decreto rilancio per il trasporto pubblico locale, sono stati stanziati 300 milioni: un terzo delle risorse potrà essere utilizzato per il ricorso a servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti e i restanti due terzi potranno essere utilizzati per coprire le perdite causate dalla riduzione dei ricavi in questi mesi di forti restrizioni. In conclusione del mio intervento, desidero evidenziare il lavoro emendativo a questo decreto-legge svolto nelle Commissioni congiunte bilancio e finanze, che ha visto concentrare l'attenzione di tutti noi su alcuni temi di interesse collettivo condivisibili e rispondenti alle esigenze dei cittadini italiani. In un momento critico come quello che stiamo vivendo, abbiamo voluto dare una risposta concreta al Paese e manterremo questa linea anche con i prossimi provvedimenti. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, insieme al senatore Presutto abbiamo deciso di seguire uno schema un po' diverso e anche un po' irrituale, rispetto al fatto di essere espressione della 5a e della 6a Commissione. Abbiamo pensato di distribuire in maniera trasversale la narrazione di quanto fosse successo, dividendo, come avete sentito dalle parole che ha appena espresso il collega, la relazione tra decreto ristori, che è l'elemento principale su cui si sono andati ad innestare gli ulteriori elementi che adesso affronteremo, e il decreto ristori due, da una parte,

su uno principale, sapendo che gli altri tre sarebbero stati fatti decadere, utilizzando lo strumento degli emendamenti da parte del Governo, era una cosa necessaria, che rispondeva oltretutto a un'urgenza. Il tema vero che ha caratterizzato la nostra azione è stato infatti quello di dare risposte rapide ed efficaci. Abbiamo pensato allora che lo strumento degli emendamenti governativi potesse essere estremamente utile per coniugare questi due aspetti: strumenti rapidi ed efficaci.

la convinzione che il Governo ha posto nel costruirlo e, dall'altra, la disponibilità dell'opposizione a ragionare privilegiando gli interessi del Paese rispetto a quelle che potevano essere contingenze politiche. È la necessità che ci porta a questo; è quello che ci circonda a indurci a questo. Ci sarà occasione in sede di replica di dettagliare in maniera più precisa e puntuale, perché adesso

ci sono i due relatori di maggioranza e le due relatrici di opposizione, ma - bene o male - abbiamo tirato tutti dalla stessa parte e, nelle notti che abbiamo passato assieme per raggiungere questo risultato, penso che con un po' di orgoglio abbiamo evidenziato come l'interesse precipuo fosse quello del Paese. Questo ci ha portato a un riconoscimento importante del lavoro dell'opposizione, che ha avuto uno sbocco anche piuttosto significativo dal punto di vista economico formale rispetto alla disponibilità assegnata al Parlamento,

Detto ciò, se questo è il quadro generale, avendo il collega ben illustrato la parte principale, ciò su cui si è andato ad innestare

sul lavoro che dovremo fare in futuro. È evidente a tutti, infatti, che non finisce qua, ma questo significa posizionarsi per costruire un percorso complesso, che penso potrà essere utile per il Paese nel suo insieme. Quindi aggredendo il tema ristori-*ter*, partiamo dal rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica per sviluppare poi il contributo a fondo perduto per i commercianti al dettaglio, alle calzature e agli accessori, passando alle misure urgenti di solidarietà alimentare, per arrivare poi all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti dal Covid-19, permettendo un incremento nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 del Fondo per le emergenze nazionali

la difficoltà - siamo sinceri - che ci siamo trovati ad affrontare nel momento in cui abbiamo approfondito questi temi. L'articolo 4 prevede l'abrogazione della facoltà di estensione degli aiuti. Vi sono poi una serie di disposizioni finanziarie piuttosto limitate limitate che, insieme all'articolo 5 (unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche), volevano rappresentare

è stato piuttosto impegnativo dal punto di vista economico, anche se gran parte di questo impegno economico si è di fatto esaurito nella proroga del termine dei versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella sospensione dei versamenti di dicembre, nella proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, nella proroga del pagamento della rottamazione-*ter*,

poi cercato di intervenire in maniera un po' più chirurgica con la razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione, così come avviene all'articolo 7, che apporta modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

il cappello che, uscendo dalla logica emergenziale, consentirà di riprendere una parte di interventi significativi che non hanno potuto avere riscontri, anche dal punto di vista emendativo (parlo sia per la maggioranza, sia per la minoranza), all'interno dei primi quattro provvedimenti.

che esca dalla logica emergenziale, per stabilire che, in maniera chiara, precisa e puntuale, Governo, maggioranza e minoranza

la parte terminale che ci permette di capire qual è stata la costruzione dell'edificio nel suo insieme e non soltanto fatto da una serie di interventi *spot*. Credo che, con questa logica, da oggi iniziamo un percorso e ringrazio tutti quelli che vi hanno collaborato con attenzione.

onorevoli colleghi, il percorso dei decreti-legge ristori è stato lungo e travagliato. Il pacchetto cosiddetto ristori è il frutto di una serie di provvedimenti che si sono susseguiti e sovrapposti negli ultimi mesi, nell'intento dichiarato di offrire sostegno alle attività duramente colpite dalla crisi economica conseguente alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid adottate dal Governo. Diversi sono i rilievi critici che possono essere sollevati, sia di metodo sia di merito. Quanto al metodo, occorre sottolineare come il modo di procedere deciso dal Governo attraverso interventi estemporanei, legati alla situazione contingente, denunci la totale assenza di una visione strategica, non tanto di lungo termine (non sarebbe comunque questo provvedimento la sede più adatta), ma nemmeno di medio termine, al punto che pochissime delle misure contenute nei quattro decreti-legge che oggi compongono il testo all'esame di questo ramo del Parlamento, adottati a poche settimane l'uno dall'altro, nel tentativo di inseguire esigenze e istanze che nel tempo sono state manifestate dalle categorie colpite dalle sempre più stringenti misure restrittive decise dal Governo, hanno un orizzonte temporale di intervento che raggiunge o supera solo i tre mesi. Questa è una modalità che, seppur possa apparire coerente con riferimento alle specifiche misure destinate al contenimento della diffusione del virus*,* mal si concilia con interventi di tipo economico e fiscale, ingenerando grave incertezza nel tessuto economico e sociale del Paese, la cui sopravvivenza è posta a serio rischio - è bene ricordarlo - dalla crisi economica più profonda dal secondo dopoguerra ad oggi. Tale modalità di procedere ha avuto inevitabili ricadute sui lavori parlamentari, che si sono svolti, anche in questa occasione, in maniera del tutto anomala, azzerando di fatto il dibattito parlamentare nelle Commissioni, proseguendo in quel percorso di esautorazione delle prerogative del Parlamento apertosi con la stagione dei DPCM e con la costituzione di una pletora di *task force* a supporto del Governo, prive di qualsivoglia legittimazione democratica, eppure così determinanti, con le loro decisioni, per la vita dei cittadini. Si sono chiesti però responsabilità e spirito di collaborazione alle opposizioni, le quali hanno tentato di dare il proprio contributo: da un lato hanno contribuito, in in alcune occasioni rivelandosi decisive al reperimento delle risorse necessarie a finanziare tutti gli interventi economici emergenziali che sono stati adottati in questi difficili mesi, attraverso l'autorizzazione dei ben quattro scostamenti di bilancio per l'anno in corso, portando l'indebitamento netto ad attestarsi al 10,4 per cento del PIL, in base alle stime del Governo, per un totale di 108,3 miliardi di indebitamento aggiuntivo autorizzato per questo esercizio finanziario. alle migliaia) sono state le proposte presentate dai Gruppi di opposizione al provvedimento in esame tese a migliorare il contenuto, senza alcun intento ostruzionistico, ma col solo obiettivo di portare sul tavolo le istanze di molte delle categorie che hanno subito maggiormente gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi sanitaria. Eppure, ancora una volta, la maggioranza si è dimostrata sorda alle nostre richieste, concedendo un ristrettissimo spazio di intervento e preoccupandosi principalmente di tenere salda la compagine di Governo. Anche con riferimento al merito del pacchetto ristori, è opportuno rilevare che diverse criticità non sono state superate non sono state superate nel passaggio parlamentare. Dal punto di vista delle risorse, si evidenzia come i primi due decreti-legge abbiano un impatto, in termini di maggior *deficit,* di circa 5 miliardi di euro per l'anno 2020; 7,8 miliardi circa è infatti la somma delle maggiori spese e delle minori entrate determinate dalle misure in essi previste, le quali trovano copertura in poco più di 2,8 miliardi di euro di minori spese, mentre l'ultimo decreto-legge approvato utilizza sostanzialmente tutti gli 8 miliardi di euro di indebitamento netto autorizzati lo scorso mese di novembre. appare interessante evidenziare, nell'analisi dei mezzi di copertura impiegati nel provvedimento in esame, è che, tra i diversi risparmi di spesa utilizzati, spiccano non solo quelli derivanti dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa legate alle diverse indennità riconosciute dal decreto-legge cura Italia, ma soprattutto quelli derivanti dal ridottissimo tiraggio del *tax credit* vacanze, misura contestata *ab origine* dalle opposizioni, ritenuta inefficace se finalizzata a dare sostegno al settore turistico-ricettivo. Non solo, ma la stessa riduzione di 5,2 miliardi di euro della dotazione del fondo destinato ad assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili della pubblica amministrazione, dimostra quanto questo Governo sia insensibile al tema della mancanza di liquidità delle imprese, affrontato attraverso lo schema dei crediti d'imposta ovvero dell'incentivazione all'indebitamento e non, come dovrebbe essere, garantendo le effettive entrate nelle casse delle aziende in difficoltà, detentrici di ingenti crediti nei confronti della pubblica amministrazione ancora insoluti. Con riferimento al contenuto delle singole misure previste, non si può invece non sottolineare come, nonostante le sollecitazioni provenienti dall'intero mondo produttivo nazionale, il Governo non sia riuscito e non abbia voluto per ora superare la logica dei codici Ateco nell'individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, generando una serie di esclusioni clamorose e ingiustificate e trovandosi a dover modificare l'allegato di volta in volta, senza del resto riuscire a trovare una soluzione che riconoscesse il ristoro - o indennizzo, come vi piace di più chiamarlo - a tutti gli operatori appartenenti alle filiere produttive coinvolte dalle chiusure. La mancata revisione dello stesso parametro di calcolo del suddetto contributo, ancorata al differenziale di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, denota ancora una volta quanto questa maggioranza sia lontana dalla realtà che stanno vivendo le piccole e medie imprese italiane. Le proroghe e le sospensioni fiscali, introdotte proprio con il decreto-legge n. 157 del 2020, sono poi arrivate in corrispondenza delle scadenze stesse, contribuendo ad aggravare la situazione di incertezza degli operatori economici, anziché cercare di diradare le nubi all'orizzonte. Emblematica è poi la proroga al 1° marzo 2021 del saldo delle rate dei piani di definizione agevolata, sospese con il decreto-legge cura Italia, prevista all'articolo 13-*ter*.4, che porrà i contribuenti che hanno attivato i piani e beneficiato della sospensione nella condizione nella condizione di dover pagare non solo le rate sospese, ma anche la rata in corso a febbraio 2021 (dunque, tre rate nello stesso mese). È stata richiesta collaborazione alle opposizioni, è stato richiesto un atteggiamento costruttivo. Da parte nostra c'è stato, ad esempio, l'emendamento 33.0.8, a prima firma della senatrice Rivolta, che riconosce alle Regioni a statuto ordinario un contributo per la riduzione del proprio debito;

siamo alla fase finale - almeno nel nostro ramo del Parlamento - di una maratona che, in un mese e mezzo, ha visto agganciarsi ben quattro decreti-legge l'uno dopo l'altro, ma che all'orizzonte vede già profilarsi il *quinquies*. Questo susseguirsi di provvedimenti evidenzia purtroppo, ancora una volta, la miopia del Governo e della maggioranza, che continuano a rincorrere il virus senza un progetto complessivo di misure serie e coraggiose a sostegno della sanità, della scuola, della cultura, dello sport e dell'economia del nostro Paese. Durante l'estate, sono mancate la prevenzione e la programmazione per la ripartenza di scuole e attività a settembre; in autunno, sono mancati gli adeguati e tempestivi sostegni per le attività economiche a seguito delle nuove restrizioni. Per un'azione efficace, in realtà, bisognava intervenire prima sullo scostamento di bilancio (pari a 8 miliardi), non il 26 novembre, e con una maggiore consistenza, così come chiesto a gran voce da Forza Italia e da tutta l'opposizione, proprio per affrontare l'urgenza. È vero che si tratta di indebitamento, ma, a questo punto e in questa situazione, è indispensabile, per non far morire i nostri artigiani, commercianti, liberi professionisti, partite IVA lavoratori autonomi, per salvare i milioni di posti di lavoro che non si salvano con il blocco dei licenziamenti, per non far morire il Paese e per cominciare a ripartire. invece, prima ha raschiato il barile, prendendo risorse qua e là e attingendo da tutti i provvedimenti - a partire dal cura Italia - risorse avanzate, perché non ben preventivate, oppure - questo è ben più grave - prese da fondi già destinati, come i 100 milioni tolti dal fondo per i ristoratori, i 5 milioni tolti dal fondo abrogato per il settore ricreativo e dell'intrattenimento o i circa 5 miliardi presi dal fondo dedicato agli enti locali per saldare, come ha ben detto la mia collega, i famosi debiti della pubblica amministrazione. Il Governo ha cercato le coperture per i decreti ristori per circa 20 miliardi dappertutto, ma non ha pensato, per esempio, di rinviare la lotteria dello scontrino, che in questo contesto storico di emergenza e crisi economica, sanitaria e sociale certamente non costituisce e non può costituire in nessun modo una priorità per il nostro Paese. Tra l'altro, oltre a prevedere importanti costi per lo Stato, anche per le assunzioni necessarie per gestire la misura, incide sulle spalle dei commercianti, per i quali solo poche centinaia di euro fanno la differenza (pensate agli ambulanti, in questo momento). Alla fine, è arrivato l'inevitabile, ma tardivo scostamento di bilancio di 8 miliardi, stanziati per finanziare buona parte del decreto-*quater*, che comprende anche una proroga delle scadenze fiscali. Peccato che tale proroga, pur attesa da tutti, sia arrivata lo stesso giorno della scadenza (il 30 novembre) e non per tutti, creando grandi scompigli per le differenti casistiche previste.

al 30 aprile per i soggetti esercenti attività rientranti negli allegati 1 e 2, inclusi i servizi di ristorazione, aventi però domicilio solo nelle Regioni rosse e arancioni. davvero incomprensibile il non aver rinviato la scadenza, per esempio, anche per i servizi di ristorazione in zona gialla, viste le restrizioni del DPCM del 25 ottobre. va detto per le scadenze tributarie e contributive del 10 dicembre, rinviate stavolta al 16 marzo, con la stessa casistica di prima, cui si aggiungono i soggetti di tutto il territorio nazionale, aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che abbiano registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020, rispetto allo stesso mese del 2019. Insomma, è un ginepraio di inclusioni ed esclusioni e di differenti scadenze, che non agevolano tutti e, di sicuro, mettono in difficoltà i liberi professionisti, a cui i contribuenti ricorrono. Vorrei sottolineare che Forza Italia, fin dall'inizio, aveva richiesto una più efficace sospensione delle scadenze fiscali, con il semestre fiscale bianco, finanche l'anno fiscale bianco, ma di certo non fatto in questo modo. Un altro ginepraio è il capitolo dei contributi a fondo perduto, che, quanto a discriminazione, non è secondo a nessuno. Con il sistema dei codici Ateco, il Governo ha messo in atto una norma che prevede contributi per alcuni (pochi) e lascia fuori interi settori, che, pur facenti parte

Per di più, l'ammontare del sostegno è calcolato come percentuale sulla differenza di fatturato del mese di aprile 2020 su aprile 2019, un criterio che non ristora con oggettività, penalizzando le attività con stagionalità sfavorevoli in quel mese. Ora però è necessario programmare da subito i provvedimenti a miglioramento e integrazione ed è impensabile proseguire sulla stessa rotta. Basti ricordare che, con il sistema della fatturazione elettronica in vigore, è immediata la lettura del fatturato e si devono considerare i costi fissi delle imprese, così come occorre modificare il sistema dei codici Ateco con la massima inclusione. Non si lasci indietro nessuno. Si proceda ad allargare anche a quelle fasce completamente dimenticate come i liberi professionisti, simpatici o antipatici che possano essere, oggetto solo del *bonus* del mese di maggio. E non si aspetti a intervenire, perché la tempistica è importante tanto quanto le risorse messe a disposizione. A tal proposito, faccio un esempio: il decreto-legge cura Italia prima il decreto-legge liquidità poi avevano previsto la possibilità di elevare il microcredito da 25.000 a 40.000 euro, liquidità importante per piccole e medie imprese, ma il problema è che tale intervento era condizionato a un decreto attuativo che non è mai stato varato (ennesima manifestazione di inefficienza burocratica, ma ormai non ci stupiamo più). L'ho anche sollecitato personalmente a più esponenti e rappresentanti del Governo,

otto lunghi mesi, in cui migliaia di micro e piccole imprese, che ricordo essere l'ossatura dell'economia italiana, sono state in attesa non di contributi a fondo perduto, ma della possibilità di contrarre debiti con cui pagare, tra l'altro, le tasse. È una cosa veramente inverosimile. Troppi oneri pesano sulle attività economiche. Anche la richiesta per la cassa integrazione prorogata di sei settimane fino al 31 gennaio 2021 comporta per molti il pagamento di un contributo addizionale, dimenticando che i datori di lavoro continuano a sostenere le spese degli istituti accessori di ogni singolo lavoratore (il TFR, i contributi previdenziali, le ferie, eccetera) e che ogni pratica per richiedere gli ammortizzatori comporta un costo. A quanto pare, però, questo Esecutivo e questa maggioranza non sanno individuare i veri problemi. Ora c'è chi pensa ad acquistare tende e a promuovere *brand* per le vaccinazioni, eppure credo che tra la Croce Rossa, l'Esercito e la Protezione civile molte strutture siano già disponibili. Questo nuovo inutile dispendioso intervento ricorda molto l'acquisto dei banchi a rotelle per la scuola; eppure la scuola non è ripartita. Cosa è stato fatto per la scuola nel decreto-legge ristori? Sono stati stanziati solo 85 milioni per la didattica a distanza: scelte che si commentano da sé, certamente deleterie per quanto incideranno sul futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. C'è poi il capitolo giustizia: Forza Italia, con tutto il centrodestra, ha messo in evidenza alcune importanti criticità sui profili di competenza della giustizia, in particolare in merito alle norme per garantire l'agibilità nella funzione giurisdizionale e il deposito degli atti, prima fra tutti quella della camera di consiglio a distanza. Come ha sottolineato più volte il senatore Caliendo in Commissione giustizia, le camere di consiglio sono essenziali per arrivare a una decisione ponderata e devono essere svolte in presenza, quindi con udienze non telematiche. Un altro aspetto su cui abbiamo insistito è stata la tutela per i magistrati onorari che si sono trovati ad affrontare l'emergenza Covid senza le necessarie coperture assicurative mediche. in tutta Italia e l'emendamento approvato dalla maggioranza; che prevede il pagamento dell'udienza anche a trattazione scritta, è assolutamente insufficiente. Un'altra criticità da noi sollevata riguarda la giustizia civile: ricordando che le competenze dei giudici di pace sono particolarmente estese, non è previsto il deposito degli atti per via telematica. Se una cancelleria è chiusa, l'utente non sa con chi interfacciarsi. Abbiamo a gran voce provato a spiegare questi problemi - ringrazio a tal proposito la senatrice Modena - per evitare queste gravi disfunzioni nel settore giustizia, ma siamo stati inascoltati L'unica apertura che il Governo e la maggioranza hanno dimostrato nei confronti dell'opposizione è stata l'accoglimento delle nostre tre proposte, su cui intervenire in maniera efficiente per il Paese: tre temi importanti, sottoscritti dall'intero centrodestra unito. la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per uso non domestico, attraverso uno sgravio sui costi fissi, con una copertura di 180 milioni di euro; la seconda il sostegno la seconda il sostegno delle convenzioni tra i Comuni e il trasporto privato con 90 milioni, una modalità che doveva essere già prevista prima; la terza riguarda un fondo di 110 milioni da assegnare alle Regioni, soprattutto quelle più colpite dal virus e quelle che, pur essendo classificate in zona gialla, hanno dovuto imporre proprie restrizioni. L'intervento su questi temi rende il nostro contributo mirato e significativo e dà un segnale chiaro sulle modalità di intervento. Certo, non siamo soddisfatti per le altre proposte non accolte e per le risorse destinate ai nostri temi, visto che ne servirebbero ben altre. Auspichiamo che in futuro, nei prossimi provvedimenti, esse possano trovare continuità anzi, consideriamo questo momento solo un preludio, per un coinvolgimento doveroso e ben più sostanzioso dell'opposizione, anche se gli ultimi segnali continuano ad essere in merito poco promettenti, come attestato dalle discussioni sul *recovery plan*, da cui è stata esclusa persino la maggioranza.

annuncia che, con il secondo *lockdown*, potrebbe arrivare al 90 per cento del fatturato. È vero che la Germania ha un'economia più solida della nostra, ma ciò dipende anche da scelte economiche e politiche fatte dai precedenti Governi. In realtà, il Governo non si deve inventare nulla, non deve avvalersi di *task force*, ma deve prendere il meglio dagli esempi virtuosi, aprendo ad un reale coinvolgimento dell'opposizione: in sintesi deve consentire al Parlamento di fare il proprio lavoro.

Signor Presidente, colleghi e componenti del Governo, c'è un solo motivo che oggi mi induce ad intervenire in discussione generale, una ragione che muove i propri passi da tempo e che troppo spesso sembra essere dimenticata in quest'Aula, che è l'eccezionalità. questa sede, nelle loro dichiarazioni fanno riferimento ai propri figli. Figli non ne ho, ma ho due splendidi nipoti adolescenti, che mi chiedono cosa sta succedendo nel Paese. Io spiego loro, con una metafora, che l'Italia, come tanti altri Paesi, è fiaccata da una malattia. Si tratta della malattia che colpisce chi viene contagiato dal Covid, ma è anche quella sorta di malattia, che colpisce il tessuto economico-produttivo, in conseguenza delle misure restrittive, adottate per contenere i contagi. Il Paese sta affrontando una gravissima malattia, che ha il volto della pandemia da Covid-19. Il Paese veste i panni di un malato a cui si devono somministrare farmaci per prepararlo ad un'operazione, che lo indeboliranno, perché devono rallentare o fermare l'avanzamento della malattia ma che gli consentiranno poi, passando attraverso una cura mirata e un'idonea riabilitazione, di tornare più forte di prima. Allo stesso modo, i provvedimenti restrittivi che abbiamo adottato per contenere la pandemia sono stati come un potentissimo antibiotico, che Presidente, sembra di stare in un bar e parliamo dei ristori.

ristori, che certo non saranno sufficienti, perché stiamo già lavorando a tante altre risposte, che andremo a dare nel prossimo anno, a partire da un ulteriore decreto-legge ristori e dal *recovery fund.* L'unica eccezionalità che veramente non si riesce a motivare è quella di una certa parte politica, seduta alla mia sinistra, che troppe volte non si sofferma sui temi in discussione.

parlato, prima, della scuola. La scuola finalmente riaprirà, il 7 gennaio, ma non lo dicono. *(Applausi)* e grazie al ministro Azzolina la scuola ha garantito, con 2,4 milioni di euro, una fornitura di arredi nelle scuole, pari a 12 volte la produzione annuale italiana. *(Commenti).* Ringraziate il ministro Azzolina

Chiedo scusa: grazie ai sindaci. Avevo sbagliato, chiedo scusa. Dinanzi a una condizione eccezionale abbiamo la responsabilità di garantire una via d'uscita a cittadini e imprese: una visione del Paese, un mosaico che si sta già progressivamente componendo. E per poterlo fare lo strumento normativo non può che essere il decreto-legge. Ricordiamoli tutti e nuovamente, anche per far capire la mole di lavoro che questo Parlamento sta responsabilmente svolgendo, supportando le misure governative che costantemente divengono sostegno e aiuto per gli italiani: cura Italia, liquidità, semplificazioni, rilancio, agosto, ristori uno, due, tre e quattro (quanti ne volete voi). con il capitolo ristori l'eccezionalità finisce per diventare anche normativa. *(Commenti)*. e vada avanti,

misure concepite per garantire ristori ai tanti settori economici contrassegnati dai cosiddetti codici Ateco, per cercare di dare risposte concrete utilizzando in modo sempre più mirato le ingenti risorse reperite nel corso del 2020,

proprio per ampliare le tutele per le attività che ricadono nelle zone rosse e arancioni e per concedere una vasta serie di proroghe alle scadenze fiscali. Quello che loro hanno chiesto, noi abbiamo fatto. Onestà intellettuale esige che si riconosca la qualità e la quantità dello sforzo profuso. Tra reindirizzamenti di fondi e il nuovo scostamento di bilancio il pacchetto ristori mette sul piatto ben 18 miliardi di euro, risorse cospicue che, tra le tante cose, ci hanno permesso di introdurre ristori fino al 400 per cento di quanto previsto dal precedente decreto rilancio, di prevedere a favore degli esercenti un *bonus* del 60 per cento per gli affitti commerciali, cedibile al proprietario...

per venire incontro alle difficoltà degli inquilini. Si prevede inoltre di cancellare la seconda rata IMU per le attività più colpite dalle restrizioni, di aumentare le mensilità coperte del reddito di emergenza, di introdurre indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo e per i lavoratori sportivi, di stanziare altri 400 milioni a beneficio dei Comuni per l'emergenza alimentare, di introdurre una vastissima serie di proroghe fiscali che riguardano Irpef, Ires, IVA, ritenute, rate di rottamazione, saldo e stralcio, di stanziare nuove risorse per le indennità delle nostre Forze dell'ordine.

e, per necessità, valuti e cerchi di realizzare una compensazione ambientale per mitigare il più possibile l'impatto negativo dell'opera. Ci stiamo avvicinando a grandi passi al Natale. A tutti noi piacerebbe farci un giro per i nostri splendidi paesi, magari prendere un caffè con i nostri cari, mangiare una pizza in pizzeria o al ristorante, farci un bagno in piscina, rilassarci in un centro termale, vederci un film al cinema o uno spettacolo a teatro. Ma non si può. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Proteggiamo i nostri affetti più cari e facciamolo specialmente con gli anziani, abbracciandoli a distanza e osservando il distanziamento fisico. Magari trascorreranno questo Natale un po' più da soli, ma credo che ne valga la pena per garantirci che nelle prossime festività avremo più possibilità di stare insieme, com'era prima di questo maledetto Covid-19. Oggi non è il momento delle becere opposizioni e del tifo da stadio per questo o per quell'emendamento, ma è il momento di andare incontro alla sofferenza dei cittadini e delle imprese. Il MoVimento 5 Stelle è immerso in questa sofferenza e intende lottare fino alla fine per portare il Paese fuori da tutto questo. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

ricordato anche oggi. Avevamo avuto una serie di assicurazioni per tutto ciò che riguardava il mondo degli autonomi e delle libere professioni,

fatto che questa maggioranza dovrebbe dimostrarci di non avere invisi gli autonomi, le partite IVA e i professionisti, ma noi ancora stiamo aspettando. *(Applausi)*. Non è stato addirittura neanche accolto un emendamento che prevedeva la sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. e più vergognosa, a mio avviso - mi dispiace molto che sia presente in Aula il sottosegretario Guerra e non il Ministro della giustizia, perché devo riconoscere che con i Sottosegretari un minimo di interlocuzione c'è stata quella di aver inserito in questo provvedimento una serie di norme delicatissime che riguardano la giustizia, che non sono state assolutamente viste, né analizzate.

abbiamo trovato invece un decreto ristori in cui questa parte è stata completamente stralciata. Alcuni miglioramenti sono passati attraverso talune componenti della maggioranza, mi pare in modo particolare da alcuni da alcuni senatori di Italia Viva, con riferimento alle questioni riguardanti l'appello e al pasticcio che è stato combinato, grazie a questo decreto, con il riesame a Milano.

anziché prendere quella norma così come era stata proposta da alcuni componenti della Commissione giustizia con il riferimento specifico, si è scritta in modo tale che oggi chiunque può avere dieci copie esecutive di un qualsiasi decreto. Voi discutete quindi degli emendamenti in cui si parla di sospensione dell'efficacia per la tutela del debitore, dopodiché fate delle norme di questo genere non capendo la conseguenza pratica,

Non sono state prese in esame neppure le proposte riferite ai giudici di pace. Mi parlate degli affollamenti, ma lo sapete che i giudici di pace hanno una competenza

vorrei la vostra attenzione su una questione. Della giustizia è stato fatto uno stralcio, stralcio, mettendo a posto quattro cose minimali. Però una cosa l'avete fatta approvare: il passaggio per fare l'esame da procuratore di Stato: mentre prima si poteva ripetere l'esame solo due volte,

oggi ci stiamo accingendo ad approvare il decreto-legge ristori e siamo tenuti a considerare attentamente le oggettive situazioni di crisi che l'Italia sta vivendo. Mi riferisco naturalmente alle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito comparti come il turismo estero, il trasporto internazionale e i consumi al dettaglio. Ma mi riferisco anche alle limitazioni che questo Governo ha imposto a determinate categorie come bar, ristoranti, alberghi, musei e spettacoli. Ora dobbiamo decidere come indennizzare, e non ristorare, chi è stato colpito duramente ed è in grave difficoltà, senza creare beneficiari di serie A e beneficiari di serie B. L'incapacità di questo Governo nella gestione della crisi si percepisce molto chiaramente, direi quasi a pelle. L'imposizione di normative non chiare ha dimostrato come la tecnica dell'improvvisazione abbia superato ogni credibile limite e, soprattutto, è la dimostrazione di come non si sia utilizzato il tempo estivo per adottare strategie, piani e metodologie di organizzazione. Personalmente, abitando in un territorio montano, la provincia di Belluno, colgo, parlando e rapportandomi con i cittadini, il sentimento e il dispiacere di come il Governo riesca ogni volta a creare situazioni di discrimine tra zone e categorie. Ancora una volta la non conoscenza del territorio si manifesta. L'Italia, nella sua diversità morfologica, determina *modus vivendi* eterogenei. Nelle zone montane, per esempio, tutti dovrebbero sapere che la gestione della quotidianità è più complessa perché il costo della vita aumenta mentre i servizi, a volte, sono ridotti all'osso o addirittura mancano. Tuttavia, noi gente di montagna resistiamo a queste difficoltà nella convinzione che abbiamo il diritto di vivere i nostri territori, le nostre tradizioni, ripagati da una genuinità sia di relazione che ambientale, aspetti che al giorno d'oggi sono raccontati sui giornali patinati o in trasmissioni televisive con narrazioni fiabesche ma senza alcuna cognizione di causa. La neve, le foto incantevoli di borghi sono realtà bellissime da vedere ma difficilissime da vivere. L'80 per cento delle persone che abita in questi territori vive grazie alla stagione turistica, soprattutto quella invernale e il fatto che il Governo, senza alcun minimo confronto né spiegazione plausibile o logica, abbia deciso di chiudere gli impianti di risalita vietare la circolazione tra Comuni i giorni di Natale e Capodanno, è stato per i cittadini un colpo complicato da incassare. Così si uccide un'economia vitale, si umilia la popolazione si accentua ancora di più il divario tra chi vive quotidianamente e chi la realtà la percepisce a volte con un certo disinteresse. Chiedo pertanto a tutti voi, colleghi della maggioranza, e al Governo di aiutarmi a dare risposte plausibili alle domande che ogni giorno raccolgo. Premetto e sottolineo mille volte che la consapevolezza che la gente di montagna ha verso la lotta al Covid è assolutamente piena. Il cuore di fiaccole della Marmolada lo dimostra. Un cuore che invito tutti a vedere perché simbolo di speranza, di vita e di salute, per la propria terra e per il proprio lavoro. Torno alle domande di cui parlavo prima: i cittadini mi chiedono perché a settembre non era rischioso far salire i ragazzi della scuola su una corriera stipata ed ora invece diventa pericolosissimo anche il trasporto di una singola persona - una alla volta - sui mezzi di mobilità del turismo invernale? *(Applausi)*. E ancora: perché la stagione estiva è stata, diciamo così, gestita in una certa maniera mentre il Governo non ha voluto nemmeno guardare i piani di sicurezza presentati dalle Regioni per il turismo invernale? Per non parlare, poi, della limitazione degli spostamenti di Natale e Capodanno tra i Comuni. L'Italia non è Roma, Milano e Napoli. L'Italia è anche piccoli centri, Comuni di 1.000 abitanti confinanti con altri Comuni che ne hanno 1.500, dove spesso abitano i componenti delle famiglie. Ma questo Governo sa come è fatto morfologicamente il Paese che dice di governare? Si direbbe proprio di no. E allora credo che sia venuto il tempo di smettere con questo atteggiamento discriminatorio, con l'arroganza gratuita e con cose che non vengono spiegate perché totalmente illogiche. Giorni fa sentivo affermare da membri del Governo, con una certa sicumera, che chiudere gli impianti di risalita equivale alla chiusura di una giostra di Luna Park. La montagna non è un Luna Park. Basta con questi paragoni così superficiali che offendono tutti, chi gestisce l'economia montana e anche chi ha un Luna Park. Non è una categoria, forse, anche chi gestisce i divertimenti? È un parlare continuo in termini di discriminazione e di non conoscenza. Preoccupatevi di capire che che questa primavera, con la mancanza di opportuni strumenti, la crisi economica si trasformerà in crisi sociale. Volete l'annientamento dell'Italia che lavora e dei cittadini che si impegnano a costruire qualcosa per loro e per lo Stato, visto che pagano le tasse. Noi montanari non siamo portati alle polemiche, tacciamo, andiamo avanti nelle difficoltà in religioso silenzio, accettiamo, abbiamo un forte senso del rispetto delle regole, ma ciò non significa che si possa prenderci per il naso come fossimo degli stupidi. Voglio anche sottolineare una certa virtuosità che ci caratterizza, portando ad esempio il fatto che durante l'estate la mia Regione, il Veneto, si è organizzata con l'aumento delle terapie intensive in forma preventiva, aumento che poi si è rivelato provvidenziale. Quello che chiediamo è di essere ascoltati, perché non c'è nulla di peggio di un sordo che non vuole sentire. Come diceva un filosofo dell'antica Grecia, la ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno, proprio l'esatto contrario di ciò che fa questo Governo con i propri cittadini e con i loro rappresentanti istituzionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, i tempi che stiamo affrontando sono complicati e le decisioni che prenderemo proietteranno i loro effetti sul futuro del nostro Paese. Il pericolo purtroppo non è ancora alle spalle, ma tanto è stato fatto e tanto altro ci accingiamo a portare a termine. L'impegno di tutti gli italiani è innegabile, lo sforzo e il sacrificio che l'emergenza ha richiesto sono stati gravosi per tutti, nessuno escluso. La scelta del nome del provvedimento non è casuale, *nomen omen.* Il decreto ristori, infatti, si pone come obiettivo quello di rifondere le categorie più colpite dalle misure di contenimento della pandemia, per risollevare anche psicologicamente tutti quei settori che più hanno patito il peso delle norme restrittive adottate con i DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre. ristori ha come missione quella di potenziare la rete di protezione intorno alle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni. I settori maggiormente interessati, oltre alla ristorazione e al suo indotto, sono stati quelli dello sport, della cultura e del turismo. L'Agenzia delle entrate ci ha recentemente certificato che tra decreto rilancio e pacchetto ristori sono stati finora effettuati più di 3 milioni di bonifici per contributi automatici a beneficio di 2,4 milioni di partite IVA, il tutto per un totale di oltre 9 miliardi di euro. Unici esclusi sono stati coloro i quali hanno attivato la partita IVA dopo il 25 ottobre 2020, per evitare possibili abusi. Quelli previsti dal decreto ristori sono aiuti consistenti e mirati che, oltre a contributi a fondo perduto, garantiscono, ad esempio, un credito di imposta per il 60 per cento degli affitti commerciali, cancellano la seconda rata dell'IMU, ampliano le settimane di cassa integrazione, prevedono proroghe dei versamenti degli acconti Irpef, Ires e IRAP per le partite IVA dei versamenti delle ritenute dell'IVA dei contributi previdenziali di dicembre per le imprese con ricavi fino a 50 milioni di euro che hanno subito una perdita di fatturato di almeno 33 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre 2019, rinvio al 10 dicembre e al 1° marzo del termine di pagamento della rata della rottamazione-*ter* e del saldo e stralcio. Il decreto ristori prevede un ulteriore aiuto per le famiglie in difficoltà, ampliando il reddito di emergenza e confermando il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021. Nel complesso, sono 18 miliardi messi a disposizione, di questi 9 miliardi sono stati reperiti grazie allo scostamento di bilancio approvato anche dalle opposizioni. Questo voto relativo allo scostamento di bilancio, che ha avuto una larga condivisione, mette in evidenza quanto in questa situazione di emergenza la collaborazione delle opposizioni sia importante e auspicabile. Mi permetto pertanto di rivolgermi alle opposizione, invitandole ad evitare di tirare fuori il peggio dello scontro politico. Rifuggiamo dai messaggi propagandistici e dalla malainformazione, non perdiamo tempo in attacchi

e improvvisare con più efficacia. Ebbene, è vero che siamo stati costretti ad improvvisare perché nessuno poteva prevedere il disastro della pandemia, una crisi sanitaria senza paragoni da affrontare con una sanità impoverita da anni di tagli e carenze strutturali, con un tessuto economico che ancora scontava

ragioni, concludo con un appello a tutte le forze politiche che siedono in quest'Aula: non sprechiamo questa occasione e dimostriamo agli italiani di essere degni del loro impegno e della resilienza che hanno dimostrato; dimostriamo con i fatti che il nostro lavoro non asseconda solo logiche di partito, ma è teso prioritariamente

Signor Presidente, Governo, colleghi, il mio intervento riprende quanto dichiarato proprio oggi dal nostro presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che dimostra ancora una volta di avere a cuore il bene dell'Italia e degli italiani prima di tutto, soprattutto e oltretutto. Nonostante infatti un Governo che fino ad oggi pare preferire le *task force* esterne alla *task force* ideale e istituzionale, che è il Parlamento, noi speriamo ancora di poter dare come opposizione seria e costruttiva e - sottolineo - opposizione, un contributo sostanziale di buon senso e utile per la tenuta e la ripresa del Paese. La linea di Forza Italia è chiarissima: lavorare dai banchi dell'opposizione nell'esclusivo interesse dell'Italia e degli italiani *(Applausi)*, confidando ancora ottimisticamente che, al di là delle ragioni di schieramento partitico, si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del Paese. Forza Italia, componente essenziale della coalizione di centrodestra, è forza di opposizione senza se e senza ma; però all'opposizione per un movimento politico come il nostro non significa assecondare gli sbagli di chi è al Governo per trarne vantaggio politico e non vorrà mai dire godere del «tanto peggio, tanto meglio» per guadagnare consenso. Al contrario, come stiamo dimostrando, come stiamo facendo come coalizione di centrodestra tutti insieme, vuol dire essere propositivi e mettersi al servizio del Paese, svolgendo il nostro ruolo con responsabilità,

almeno con la magra soddisfazione, per il momento, di dimostrare cosa faremmo praticamente se fossimo noi a poter decidere. In questo momento storico

come contropartita solamente di veder accolte quelle proposte di buonsenso e di visione, come il ristoro dei costi fissi delle aziende e delle attività produttive o l'anno bianco fiscale, promesso proprio in questi giorni dal ministro Di Maio, in risposta alle nostre sollecitazioni. Amen, così sia, perché le nostre piccole e medie imprese, le nostre realtà produttive, le attività di servizio, come gli eventi, i matrimoni, i commercianti, gli artigiani, gli ambulanti, il settore edile e i trasportatori privati, hanno bisogno di sostegno certo e di speranza nel futuro per non mollare. Tale speranza può darla solo un Governo capace, competente e lungimirante, che non si limita a mettere pezze sui buchi mano a mano che si formano. I sacrifici si possono chiedere se si è in grado di dare sicurezza, non senza certezze. Ci sono poi i giovani e, con loro, il sostegno alla scuola e al lavoro. Ringraziamo il ministro Azzolina, caro senatore Santillo, per la miseria degli 85 milioni destinati alla didattica a distanza, per gli inutili banchi a rotelle per cui si sono buttati via i banchi nuovi. *(Applausi)*. La ringraziamo anche per i ragazzi disabili lasciati senza gli insegnanti di sostegno e per la richiusura quasi immediata delle scuole subito dopo la riapertura estiva per non aver pensato a cose semplici, come il doppio turno di entrata e la convenzione tra trasporto pubblico e trasporto privato. Avrebbe almeno dovuto parlare con il ministro De Micheli, evitandole la brutta figura di proporre la scuola aperta la domenica o la negazione che il virus possa girare sui mezzi di trasporto. Serve intelligenza, perché non vorremmo mai parlare di una generazione Covid. Servono inoltre risorse consistenti, volontà politica per riqualificare l'istruzione, quella tecnica superiore e la digitalizzazione e, soprattutto, interventi mirati per la vera, coraggiosa, rivoluzione della scuola: la garanzia della libertà di scelta educativa. *(Applausi)*. Infatti, la libertà di scelta educativa è quella che fa di un Paese un grande Paese e si realizza solo attraverso il sostegno paritetico alla scuola statale e alla scuola paritaria. La scuola paritaria è la grande dimenticata di questa crisi. Peraltro, parlare di dimenticanza non è corretto, parliamo di un vero e proprio disegno di una parte della maggioranza - il MoVimento 5 Stelle - con la complicità della restante parte - la sinistra - che continua a peccare per omissione di intervento. Vi sono grandi proclami di volontà,

centrodestra: la concessione di fondi alle Regioni più colpite dal Covid (che ci sembra un emendamento di grande buon senso); la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese; un maggior sostegno al trasporto locale.

Lavoreremo di concerto con l'iniziativa privata, quella che a voi fa tanta paura e tanto timore, a ogni livello. Il nostro obiettivo è che lo Stato e l'impresa lavorino insieme. Lo Stato deve imparare dalle imprese, che si sono rivelate bravissime comunque, nonostante voi, a tenere botta a questo momento di crisi, da alleati e non da antagonisti. quindi chiediamo alleanza tra Stato e impresa, tra Stato e lavoratori, tra Stato e famiglia, tra Stato e scuola, affinché i cittadini abbiano ben chiaro che il nemico è là fuori e si chiama Covid e crisi. Il nemico non può certo essere lo Stato, il Governo. Avremmo Governo. Avremmo voluto fare molte cose. Penso, per esempio, ai sindaci che mi hanno chiesto di avere fondi per aiutare i cittadini non soltanto

perché la gente non ce la fa più ad alzarsi al mattino non sapendo oggi cosa dovrà fare domani e avere chiari adempimenti e scadenze. Lasciateci liberi, lasciate libere le imprese.

purtroppo non bastano piccole aperture solo in quest'Aula e qualche concessione fatta a noi dell'opposizione, tra l'altro strappata non senza fatica questo ringrazio la nostra relatrice, la collega Ferrero, che è anche Capogruppo in Commissione bilancio - per poter finalmente parlare di collaborazione tra maggioranza e opposizione. La crisi che viviamo si supera con atti concreti, tangibili, che non lasciano davvero nessuno indietro. In mano a questo Governo i decreti-legge sono degli ossimori, la certificazione dell'incapacità della vostra politica di dare risposte agli italiani e, cioè esattamente il contrario di quello che dovreste fare.

Si parla dei comportamenti irresponsabili dei cittadini, ma responsabili devono essere prima di tutto coloro che emanano i provvedimenti, e cioè voi che governate questo Paese. Dovreste interrogarvi un po' di più sulla morte economica più grave, quella del commercio, quella del turismo, quella della ristorazione.

chi fa lo stesso servizio con *bus* scoperti, solo perché ha una dicitura fiscale diversa. Questa per noi è non una misura di ristoro, ma una marchetta! Vergognatevi! In Italia decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare stanno subendo i contraccolpi della crisi economica causata da un'epidemia che voi non siete assolutamente capaci di contrastare in alcun modo. Eppure - come abbiamo già detto - l'agroalimentare vale 210 miliardi di euro, ma ricordiamoci che nel fuori casa è calato del 48 per cento, con una perdita complessiva sull'agroalimentare e sulla spesa alimentare di oltre 41 miliardi di euro.

la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari per 3,5 miliardi e riguarderà soprattutto vino e ortofrutta fresca e trasformata; un danno enorme che dovrebbe essere compensato dall'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese.

che stanziava 100 milioni di euro per le filiere agroalimentari che sono fondamentali, importantissime: penso alla zootecnia, al problema attuale della suinicoltura, al latte, all'apicoltura, al florovivaismo, al vino. prevedeva un meccanismo di sostegno forte e vero all'agroalimentare italiano. Parliamo di *made in Italy* e poi ci nascondiamo dietro un dito e togliamo le risorse per darle, magari, a un assistenzialismo forzato che non genera occupazione. per i nostri contadini, per i nostri agricoltori - 100 milioni di euro per la cambiale agraria, 30.000 euro per ogni azienda: a dieci anni avrebbero restituito quelle risorse a tasso zero.

abbiamo chiesto la semplificazione sul percepimento dei fondi europei, la PAC, per le aziende. Oggi per avere un certificato antimafia dalle prefetture che lavorano in *smart working* ci vogliono mesi, e, se manca quello, non arrivano le risorse, e fa liquidità. Abbiamo chiesto 600 euro di *bonus* per ogni piccolo agricoltore e contadino

Cari colleghi, ci avviciniamo al santo Natale. Gli italiani tutto vorrebbero trovare sotto l'albero tranne i pacchi del Governo: l'aumento esponenziale del debito pubblico...

gli italiani non vogliono trovare il pacco del Governo sotto l'albero: l'aumento esponenziale del debito pubblico, l'aumento della disoccupazione, precarietà, scuole chiuse da mesi, anziani soli, enti locali abbandonati. Fate un bel regalo lo dica ai Ministri di questo Governo - a tutti gli italiani: andate a casa e cercatevi un lavoro degno delle vostre capacità, che vi chiediamo di togliere al servizio del Paese, perché altrimenti non ci rialzeremo mai più. Prima gli italiani, sempre. *(Applausi).* È iscritto a parlare il senatore Anastasi. Ne ha facoltà. con un nuovo decreto-legge ristori - il quarto in poco più di un mese - continua e si estende ulteriormente l'azione del nostro Governo a sostegno dei lavoratori, dei professionisti, delle imprese e delle famiglie italiane. L'intero pacchetto ristori si presenta oggi all'attenzione di quest'Assemblea con importanti correttivi: una vasta serie di proroghe fiscali e misure ristorative, fra le quali degne di menzione sono i rimborsi per i proprietari di immobili che concederanno sconti sugli affitti; una norma sperimentale - come l'ha definita il presidente Pesco - per andare incontro alle esigenze di chi è in locazione e magari sta affrontando mille difficoltà; una misura che permette una riduzione del canone, limitando l'onere per il proprietario. Sempre a firma del presidente Pesco è l'emendamento pensato per sostenere famiglie e imprese indebitate, che anticipa alcune misure sul fallimento e le crisi d'azienda. Merita di essere menzionata anche l'iniziativa dello stesso collega sulla proroga del cosiddetto fondo Gasparrini. Altrettanto significativo è l'emendamento del senatore Romano, con cui si stabilisce che non subiranno prelievo fiscale le imprese e i professionisti che hanno ricevuto dallo Stato contributi, indennità e e *bonus* contro la crisi Covid-19. Abbiamo approvato persino un emendamento non di maggioranza sull'equo compenso per le consulenze e le prestazioni professionali sul superbonus 110 per cento - finalmente anche l'opposizione si accorge della nostra eccellente misura e uno sul fondo dedicato al pagamento delle bollette per imprese e professionisti, come già il Governo aveva legiferato nel decreto-legge liquidità, dimostrando con i fatti che le proposte di buonsenso da noi trovano accoglienza

per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico-produttivo. Ed è con questo spirito che continueremo ad avanzare idee e proposte. Un ultimo appunto è sull'emendamento che non c'è. Avevamo posto in questo decreto all'attenzione di Governo e Parlamento l'estensione del superbonus 110 per cento. Poiché tutti a parole dicono di volere la proroga, ma nei fatti non vi è ancora alcuna risposta in merito, invito la maggioranza di Governo a trovare il coraggio di fare la cosa giusta. Sono tempi eccezionali. La storia ci giudicherà per cosa abbiamo fatto e non per le buone intenzioni e le belle parole. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli senatori, il percorso politico di questi decreti-legge che veniamo a discutere è stato complesso, ma il Paese e il Parlamento ne hanno recepito la necessità e l'importanza. Ritengo, dunque, che giungere alla loro conversione in legge rappresenti un significativo punto di partenza e ripartenza per tutti noi. Vorrei dire allora che dobbiamo trarre profitto da questa discussione, coglierla come l'occasione che abbiamo cercato per ricollegarsi alle nostre comunità, essendo parte del rapporto armonico tra la *polis* e gli individui che la compongono. La fatica di questa composizione è l'obbligo che ci siamo assunti quando abbiamo accettato di rappresentare tutto il popolo come singoli senatori e come Assemblea. La pandemia ha colpito e incrinato indistintamente il cosmo della civiltà, in particolare quella occidentale, suscitando il senso della nostra umana inadeguatezza, sovvertendo molti punti di riferimento che davamo per acquisiti. Ci si è sgretolato in mano il mito asettico del progresso scientifico infinito e invincibile; è caduto il velo dell'illusione di essere cloni del pericoloso modello di Übermensch futuribile. In un colpo solo, salute, ambiente, economia, protezione sociale rapporti internazionali sono apparsi un tutt'uno indissolubile, e di questo dobbiamo farci carico. La pandemia ci ha fatto anche intendere senza ombra di dubbio quanto reale sia questa nuova forma di isonomia, l'uguaglianza di fronte al rischio che tutti i cittadini indistintamente corrono di essere travolti dal virus. Siamo anche stati messi di fronte a spaventevoli, per quanto ipotetiche, classificazioni di gerarchie legate all'età o a situazioni di salute correlate all'accesso alle cure. Ora, l'appello del Presidente della Repubblica a ritrovare l'unità per costruire la risposta adeguata che il Paese ci chiede è stato colto e raccolto per darci l'opportunità di mantenere una dignità che la Costituzione garantisce come fondamento imprescindibile. Sono stati e saranno ancora mesi lunghi e difficili e questi ristori rappresentano un impulso a rinnovare la fede comune sul valore che i Padri costituenti hanno inciso alle fondamenta: l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e ora più che mai il lavoro e la dignità dei lavoratori dobbiamo tutelare e sostenere. Trovare un linguaggio comune durante i lavori delle Commissioni congiunte; ridimensionare la mole delle migliaia di emendamenti su cui maggioranza e opposizione hanno lavorato; trovare la quadra su quanto il Governo potrà fare per la nostra comunità nazionale sono stati per tutti difficili e impegnativi. Ristorare rappresenta, dunque, un passaggio politico di alto valore democratico, ma soprattutto un segnale forte e inequivocabile che si vuole ripartire dai cittadini, dalle peculiari necessità di chi è stato in vario modo colpito. Chi ha voluto speculare sulle possibilità di mettere in difficoltà il Governo ha fatto un gioco spregiudicato in primo luogo verso i cittadini. Invece, mai come ora, dobbiamo renderci conto che le risorse dei decreti messi a disposizione con i ristori del Governo e con la volontà politica della maggioranza rappresentano un impegno di portata straordinaria per l'intera comunità nazionale. Sono risorse indispensabili per tamponare i bisogni da una parte, ma soprattutto per porre le basi di un disegno nuovo e più complesso che verrà definito nei prossimi mesi con il Next generation EU, e che dovrà necessariamente coinvolgere tutte le istituzioni, il Parlamento, così come le Regioni e gli enti locali o le realtà specifiche, e permetterci di rifondere una prospettiva di futuro che la pandemia ha drammaticamente interrotto. Molti sono stati i capitoli, molte le problematiche affrontate durante le audizioni e la discussione. Tra le varie e innumerevoli misure avviate mi preme rivolgere un'attenzione particolare a due complessità, che sono parte integrante della realtà italiana e hanno estremo bisogno di essere sostenute. Abbiamo sempre asserito quanto sia importante in questo momento non dimenticare i più deboli: tra questi i soggetti più esposti sono le persone con disabilità o malattie disabilitanti e le loro famiglie, che non devono in alcun modo essere lasciate sole. Il Covid, infatti, ha ridotto la possibilità di aiuto e intervento alle famiglie. Si devono dunque aumentare le risorse e il numero delle residenze socio-assistenziali; aumentare l'impegno per progetti individuali e moduli respiro, perché la disabilità è una condizione di vita, e non uno stato temporale. La malattia degli operatori ha contribuito a ridurre i servizi delle residenze, anche quelle protette per anziani o i malati cronici. E non ci siamo dimenticati dei genitori anziani degli utenti delle residenze socioassistenziali, che risultano ad alto rischio di contagio e fortemente preoccupati per il futuro dei loro figli, oltre che per se stessi. Il secondo tema riguarda la cultura, a cui abbiamo cercato di dare massima attenzione. Ci sono categorie di lavoratori che stanno vivendo questa crisi pandemica in modo drammatico. C'è stato qualcuno che ha asserito come con la cultura non si mangi, ma il nostro è un Paese che vive di cultura e viene riconosciuto nel mondo anche per la cultura. I lavoratori dello spettacolo, tra cui attori, musicisti e i cosiddetti lavoratori intermittenti, ma anche studiosi e ricercatori nel campo umanistico, traduttori, sono categorie determinanti e di formazione altissima che non vengono considerate da molti come parte produttiva del Paese. Al contrario, come scrive Claudio Magris nel suo accorato appello sul «Corriere della Sera», sono professionisti appassionati e altamente qualificati che spesso vivono di contratti occasionali e precari con teatri, fondazioni, istituzioni, atenei e case editrici. L'impegno che ci muove è di ritrovare la centralità di queste categorie per evitare il grave declino di un'eccellenza che ci identifica e ci qualifica nei confronti dell'Europa e del mondo intero.

Devo essere sincero: se vogliamo parlare agli italiani con le parole chiare, sicuramente non lo possiamo fare se non facciamo delle norme chiare. Sfido voi

Su questo punto, facendo parte della Commissione giustizia, non posso che ricollegarmi, sottoscrivendole, alle dichiarazioni già rese dalla senatrice Modena in materia di giustizia. Voi avete inserito all'interno di un decreto-legge di natura economica delle norme in materia di giustizia assolutamente folli, perché non si può pensare di normare la giustizia sotto l'egida del Ministero dell'economia e delle finanze. Anzi, nel ringraziare il sottosegretario Guerra,

dunque alla maggioranza di smettere di governare con falso buon senso, perché - citando Guareschi - state governando non con buon senso, ma semplicemente con senso comune, che è molto peggio. Rischiate dunque di fare dei danni clamorosi.

«Fai il *bonus* vacanze e poi *te 'ncazzi* che la gente va in vacanza, fai il *cashback* di Natale e poi *te 'ncazzi* se la gente va a fare acquisti» *(Applausi)*: se questo è il modo di fare politica della maggioranza, evidentemente è il momento di andare a casa. Buon Natale!

alcuni locali pubblici, come è successo in Sardegna, in cui società *offshore* sono state favorite, lasciando affollare le loro discoteche, a discapito della salute di tutti. Il preavviso ci è stato dato da diversi Paesi europei, dove già a settembre si contavano i nuovi contagi a decine di migliaia al giorno. In Italia l'impennata si è palesata a ottobre, così che il 7 ottobre si è reso necessario prorogare i termini dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Da quel momento in poi, con il crescere del numero dei contagi, è stato un susseguirsi di DPCM e decreti-legge per contrastare la diffusione del virus, confermando la pressione sugli ospedali e inevitabilmente adottando misure sempre più restrittive, fino ad arrivare alla suddivisione per aree di maggiore o minore contagio a carattere regionale. Il decreto-legge ristori del 28 ottobre ha avviato una serie di altri decreti-legge, visto il proseguire dei contagi, per stanziare risorse a fondo perduto e agevolazioni fiscali ed economiche per le attività colpite dalle necessarie Fra le misure principali rileviamo il contributo a fondo perduto per le partite IVA (ampliando i settori di intervento rispetto ai beneficiari individuati dal decreto rilancio); proroga della cassa integrazione (altre sei settimane da usufruire tra il 16 novembre e il 31 gennaio); il credito d'imposta per gli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata IMU; l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello sport e dello spettacolo; la nuova *tranche* del reddito di emergenza. Insomma, con i decreti ristori fin qui emanati abbiamo stanziato per le attività colpite circa 19 miliardi di euro, mentre altre risorse stanno per essere stanziate nell'imminente legge di bilancio. In questi mesi l'agricoltura non è stata trascurata. Sono stati stanziati 4 miliardi per il settore, e di questi un miliardo è destinato all'esonero contributivo per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca

il supporto economico alle attività turistiche e della ristorazione situate nelle aree protette; il credito di imposta per gli aumenti di capitale; le garanzie per la liquidità delle imprese agricole e della pesca; i contributi a fondo perduto e i mutui a tasso zero in favore delle aziende agricole. E ancora: il fondo per le emergenze alimentari; il contrasto allo spreco; il fondo ristorazione per sostenere il *made in Italy*; il sostegno all'imprenditoria femminile con il progetto "Donne in campo"; il sostegno all'occupazione giovanile in agricoltura. Su queste e altre misure verranno stanziate altre risorse nella legge di bilancio. Per il settore primario siamo a un punto cruciale. Grande è il suo ruolo in termini di *export*, nuova PAC, *green new deal*,con le strategie *farm to fork* e l'incremento del biologico; un settore in cui possiamo vantare primati e attenzione alle problematiche in misura maggiore e migliore rispetto agli altri Paesi. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza dobbiamo mettere mano alla competitività del sistema alimentare, con l'ammodernamento dei sistemi produttivi orientato alla sostenibilità; la prevenzione del dissesto idrogeologico e il rafforzamento dell'agrosistema irriguo; la gestione forestale sostenibile e il recupero delle aree rurali abbandonate. Sono queste le sfide che ci apprestiamo ad affrontare e lo stiamo facendo con tutta l'accortezza che necessita. Ma il lavoro viene meglio con la condivisione di responsabilità e impegno da parte di tutti. La rapidità e l'efficacia con cui sono state trovate le risorse per compensare almeno in parte le mancate entrate delle attività economiche hanno ancora una volta dimostrato l'attenzione che questo Governo, insieme al Parlamento, riversando verso una pandemia che sta cambiando paradigmi e visioni in ogni situazione a livello planetario. In questo sciagurato periodo, che ormai va avanti da circa un anno, in tutte le occasioni non si è mai mancato di sottolineare come la collaborazione politico-istituzionale, oltre che di tutte le attività private e dei cittadini, fosse assolutamente necessaria per arrivare al traguardo dell'uscita definitiva dall'emergenza causata dalla pandemia. Non ci stanchiamo di ribadire questo concetto, poiché tutte le manifestazioni di disinteresse o di vacua polemica non faranno altro che porre ulteriori ostacoli al raggiungimento del risultato. Inoltre, ci tengo a sottolineare che non è più possibile abbassare la guardia sulla prevenzione. È indispensabile incrementare gli sforzi per contrastare eventuali nuove evoluzioni di virus di varia provenienza attraverso il rafforzamento della ricerca scientifica. è essenziale il miglioramento delle strutture sanitarie presenti sul territorio italiano, che hanno mostrato in modo evidente grossi limiti derivati dai tagli e dalla mala gestione degli ultimi anni. ristori in esame deve essere il trampolino di lancio verso una nuova visione di economia, di sviluppo e di lavoro, quella che finora non c'è stata, e i risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti. Questo Governo sta dando una svolta al sistema che ha logorato la nostra bella Italia, aiutando tutti a rialzarsi

peraltro dati ad alcuni mentre altri sono stati completamente dimenticati: lo hanno detto i miei colleghi prima ed è inutile che lo ribadisca. Il mio intervento sarà limitato a un settore ben preciso - come ha detto prima la senatrice Modena decreti-legge in questione, con ben dieci - anzi, di più - articoli, ma che è stato completamente ignorato nella Commissione di merito attraverso un passaggio quasi da fuggitivo della situazione, cioè tutto il tema giustizia. In un momento di emergenza e in uno stato di eccezione, qual è quello che stiamo vivendo, conseguente alla pandemia e che qualcuno ha definito una vera una vera e propria situazione bellica, il tema giustizia reca con sé dei paradigmi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti penali e il processo penale, che non sono trascurabili.

e con il suo articolo 83 abbiamo introdotto dei principi dovuti all'esigenza e al momento, e cioè il fatto che le udienze si

irrompe sulla scena un altro principio. In base ad esso addirittura il processo penale di secondo grado, tolta l'ipotesi della rinnovazione dibattimentale, diventa un processo cartolare: il pubblico ministero fa l'appello, la difesa non c'è mai stata in primo grado e presenta delle conclusioni scritte - se arrivano, perché non si sa in che modo ai giudizi riuniti in camera di consiglio; anzi, non sono riuniti simultaneamente, ma ognuno dal proprio ufficio, ognuno dalla propria residenza e attraverso una riunione simbolica. Ecco, ciò significa dematerializzare, perché si è inteso in tal modo modo affrontare un'emergenza. Questo certamente è comprensibile, ma noi lo avremmo compreso nella misura in cui tutto ciò serva ad agevolare l'attività degli operatori del diritto. Tutto ciò l'avremmo compreso nella misura in cui non ci siano norme incongruenti tipo quella del 415-*bis* del codice di procedura penale,

certamente certificata dai sistemi del Ministero. Che cosa cambia? Cambia l'epistemologia giudiziaria, e cioè la concezione stessa del processo. cambia in modo pericoloso perché, se a un processo che si svolge nella parità, nel contraddittorio della formazione della prova tra due parti uguali, noi togliamo ad una di esse, che normalmente è minoritaria nell'esercizio dei poteri, ossia la parte della difesa, il proscenio, la possibilità di esercitarsi e di esercitare le sue funzioni davanti a un giudice terzo, abbiamo ucciso il processo penale. Questo è evidente e si rifletterà. Se quello è l'indirizzo che volete imprimere all'era *post* Covid - e ci auguriamo tutti che l'emergenza finisca realmente, secondo quanto dice questo decreto, il 31 gennaio 2021 - mi chiedo quali e quante norme saranno in vigore allora, perché non abbiamo già oggi l'esatta contezza di quali norme saranno applicabili nel momento in cui la pandemia sarà superata.

Il processo civile in Italia dura tremila giorni, oltre il doppio di quanto accade mediamente nei Paesi europei. E questo produce - secondo statistiche riconosciute da tutti - un danno di circa tre miliardi per le imprese e e un mancato guadagno, in termini di investimento, di circa 11 miliardi nel nostro Paese. Vogliamo capire che, se le idee camminano sulle gambe degli uomini, così anche la giustizia non può che camminare sulle gambe degli uomini? Abbiamo bisogno

molto chiaro, anche perché ultimamente ho ascoltato alcuni interventi in Commissione dei vari Sottosegretari che cortesemente hanno risposto alle nostre interrogazioni. Poi c'è una questione di fondo, secondo me costituzionale, che non è stata esplorata in modo opportuno. Noi sappiamo che l'articolo 111 della Costituzione riserva l'attuazione del giusto processo alla legge, e cioè contiene un'espressa riserva di legge. In realtà, nel momento in cui,

che lo svolgimento del processo penale viene regolato dal deposito degli atti, ferme restando le garanzie processuali, attraverso un regolamento del responsabile del Ministero

dei Radicali e di Rita Bernardini che stanno denunciando la situazione delle carceri in Italia. Vorrei che il Ministro, una volta tanto, desse i numeri. Sappiamo purtroppo che è una sua specialità quella di dare i numeri, perché abbiamo visto che cosa è riuscito a fare con la prescrizione. *(Applausi)*. Abbiamo visto che cosa è riuscito a fare con il cosiddetto spazzacorrotti. Ma vorremmo che desse realmente i numeri della situazione carceraria in Italia. C'è un sovraffollamento di oltre 4.000 detenuti. Qual è la situazione delle carceri oggi? Ci sono circa 1.000 detenuti affetti da Covid, oltre 500 agenti

Io non so cosa sarà: immagino che sia molto difficile rimettere insieme e pensare al sistema delle pene in Italia dopo quello che è successo, anche perché probabilmente la nostra capacità di reagire rispetto a quanto sta accadendo poggia su basi abbastanza fragili anzi,

che ha un obiettivo, quello di porre rimedio a un'ingiustizia nei confronti di coloro che non si devono solo chiamare eroi, ma devono essere tutelati concretamente vale a dire medici, infermieri, in generale operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Covid. Nonostante gli stanziamenti multimiliardari, non si sono trovati 100 milioni di euro per sostenere questo tipo di bisogni e tutto questo in uno scenario che è assolutamente in contrasto con i fondamentali della dignità e dell'etica. Ebbene, in questo contesto è di tutta evidenza che troppo spesso si è fatto riferimento a parole che hanno trovato il loro fondamento e la loro attenzione in un processo di condivisione tale per cui

per alcuni di loro, a mio modo di vedere ancor più grave, posto che

facendo valere chissà quale codicillo sottoscritto tra clausole vessatorie, sul presupposto che l'infezione da Covid non rientrerebbe nell'ambito del concetto di infortunio, ma in quello di malattia, distinguendo tra causa violenta e causa virulenta. Abbiamo aderito al processo di integrazione normativa con il testo base n. 1894 in 1a Commissione in sede redigente, in previsione

però l'opportunità della conversione dei decreti ristori, abbiamo ritenuto di promuovere ben tre emendamenti sull'argomento, che avrebbero anticipato le misure di ristoro economico non ulteriormente rimandabili, dal nostro punto di vista, stati inspiegabilmente rigettati, negando addirittura l'approvazione in termini di impegno

disattendere anche su argomenti così sensibili da rendere inaccettabile la democratura a cui state cercando di abituare il Paese,

più che ristori elargisce elemosine ad alcuni settori colpiti dalla seconda ondata, che questo Governo ha saputo soltanto annunciare, ma non gestire. Sul punto bisognerebbe fare chiarezza.

ossia che, se oggi ne parliamo e siamo costretti a investire le risorse del quarto scostamento di bilancio, è per colpa di un Governo che non è stato capace di impedire che la seconda ondata si abbattesse con violenza sull'intero Paese. Nel solco di questa stessa logica, che possiamo dire più che approssimativa, si muove il decreto-legge, continuando a seguire un profilo emergenziale, senza affrontare nel merito le difficoltà di chi è rimasto indietro a causa della crisi economica. Le attività si aspettavano infatti da parte dello Stato non elargizioni, ma interventi coraggiosi, come rinuncia alle proprie pretese. Si è invece proceduto con sospensione o dilazione di imposte, con la diretta conseguenza che, se non vi saranno manovre massicce e importanti a sostegno dell'economia, le attività che a fatica sono rimaste in piedi nel 2021 e nel 2022 si troveranno strangolate dalle scadenze di oggi e anche di domani. Con la nostra *leader* Giorgia Meloni abbiamo tenuto una conferenza stampa nella quale abbiamo presentato il decreto ristori, proponendo serie e concrete proposte per abbattere la crisi economica, ribadendo soprattutto che non è quella del sussidio, a cui purtroppo alcuni partiti della maggioranza (e mi riferisco al MoVimento 5 Stelle) sono affezionati, ma quella di seguire l'abbattimento dei costi fissi. Sono questi oggi a rappresentare il maggiore ostacolo per tantissimi imprenditori e anche professionisti, grandi e piccoli, per uscire da questa crisi che attanaglia tutti. Sul punto avreste dovuto concentrare la vostra attenzione, piuttosto che continuare nella logica degli interventi a pioggia. Ugualmente, avreste dovuto correggere gli errori sulle tempistiche che già nei precedenti provvedimenti si erano dimostrate inadeguate. Le casse integrazioni sono arrivate con estremo ritardo e la maggior parte degli imprenditori ha dovuto anticipare di tasca propria o si è trovata costretta anche a sostenere le spese delle liquidazioni di coloro che hanno preferito cercare un'opportunità lavorativa altrove. Ciò non solo perché i vari decreti ristori, come nel caso, appunto, ricettivo, hanno la loro base in fondamenta errate o quantomeno sottostimate, cioè la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020: è possibile che dietro questa scelta ci sia

ottenuti (quando arrivati) bastano appena a coprire una piccola parte fissa delle imposte. E per vivere? Sarebbe piuttosto stato opportuno, volendo ragionare in un'ottica

ricettivo non è che uno dei tanti settori che lamentano l'inadeguatezza di questo provvedimento, in quanto ce ne sono molti altri che denunciano il completo abbandono da parte del Governo. Ad esempio, cosa è stato fatto per il settore turistico? Oggi non prevedete alcun ristoro o misure di sostegno adeguate. Inoltre, avete completamente dimenticato le agenzie di viaggio, una categoria completamente messa in un angolo con un codice Ateco

che queste attività possano andare avanti, se in dieci mesi nulla è stato ancora fatto e nulla hanno ancora ricevuto? Le agenzie di viaggio sono oltre 10.000 in tutta Italia e occupano migliaia di persone, con un risultato molto impattante sul nostro PIL. Occorre inoltre considerare che la paura, che continua a farla da padrone, difficilmente consentirà di tornare subito a viaggiare come La stessa domanda potremmo farla per il settore degli eventi, visto che sono stati cancellati più del 90 per cento degli eventi culturali e religiosi. Nel 2020 matrimoni, comunioni, concerti, sfilate di moda e spettacoli sono stati completamente annullati. Si tratta di un mondo intero che da quasi un anno è fermo e di centinaia di migliaia di professionisti impegnati in questa attività o nel loro indotto che hanno percepito poco o quasi nulla. impegnati nella ristorazione, come bar e ristoranti. Qui il Governo ha fatto ancora peggio, obbligandoli a investire risorse in presidi igienico-sanitari e a ridurre i posti a sedere, sacrificando anche licenziati) e imponendo l'acquisto di ulteriori *dehor*. Poi che avete fatto? Li avete di fatto chiusi o ridotti in maniera drammatica nella loro offerta di servizi, imponendo loro anche una chiusura alle ore considerare che si erano organizzati, riuscendo a garantire il servizio in condizioni di sicurezza. Non avete fatto alcuna distinzione: per voi sono diventati

unitamente alle norme di igiene, che sono diventate patrimonio del nostro comportamento quotidiano? Inspiegabile, poi, che alcune attività legate al settore dell'artigianato siano state dimenticate, così come avvenuto per i servizi alle persone. Che dire degli ambulanti, cui avete imposto il divieto di

benissimo e vi assicuro che non vi è la possibilità di assembramento; ciononostante, lo avete chiuso, con la conseguenza che lentamente le attività che lavorano al suo interno andranno a morire. Si tratta quindi di un'agonia lenta. Un altro tema sul quale il decreto-legge avrebbe dovuto prevedere un intervento è quello dei finanziamenti, anche garantiti, per le imprese ricettive. Oggi queste attività sono considerate a rischio, quindi non vengono erogati finanziamenti, nemmeno quelli garantiti al 90 per cento dallo Stato; per questo motivo, sarebbe necessario prevedere un allungamento almeno a vent'anni dei prestiti garantiti al 100 per cento dallo Stato e l'incremento anche a importi ben superiori degli odierni 30.000 euro, senza che le imprese vengano sottoposte a revisione del merito creditizio.

in esame Fratelli d'Italia ha confermato quella serietà e quella concretezza che sono state l'elemento determinante della nostra crescita di consenso tra gli elettori. Infatti, è stato approvato un nostro emendamento volto a potenziare il trasporto pubblico locale; sicuramente è importante, ma da questo momento Regioni e Comuni potranno anche stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenze per per l'esercizio di taxi e per i noleggi con conducente (NCC). Da tempo Fratelli d'Italia ripete che la soluzione non è vietare e chiudere, quanto piuttosto adeguare la nostra offerta di servizi alla nuova situazione. È noto che i trasporti rappresentano la vera falla del sistema, alla quale il Governo e la maggioranza non sono stati capaci di opporre valide soluzioni. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, dicendo che il limite della capienza rappresenta sicuramente un numero senza senso, perché mancano i controlli; un potenziamento dell'offerta di servizio, come diciamo dall'inizio della pandemia, per ridurre l'afflusso. Sarebbero opportuni più ascolto e meno arroganza, più condivisione e meno dirette *streaming.* Di questo hanno bisogno gli italiani, in questo difficile momento.

voglio la libertà che mi avete sottratto. Queste sono le parole del signor Carlo Gilardi, novantenne di Airuno, un piccolo paese di della provincia di Lecco, ci viene raccontata in questi giorni dalla nota trasmissione televisiva «Le iene». È la storia di un anziano, membro di una famiglia decisamente benestante, un uomo decisamente di cultura e decisamente generoso. La sua generosità lo ha reso famoso nel suo piccolo Comune, non soltanto per i gesti di altruismo verso singole persone e intere famiglie, ma perché anche il Comune in cui abita si è giovato delle sue azioni: ha avuto in donazione un defibrillatore;

a seguito di un esposto del signor Carlo, in cui venivano riportati episodi gravissimi, come l'emissione di vaglia dell'amministratore delegato verso amici, senza una giusta causa.

La vita del signor Carlo potrebbe somigliare a quella di San Francesco. Immaginiamo quale storia potremmo raccontare oggi e quale sarebbe stata la vita di San Francesco ai tempi dell'amministrazione di sostegno. Avviandomi alla conclusione, vorrei dire una cosa da questo scranno:

in questa vicenda sono state decisive per la vita del signor Carlo, che oggi è rinchiuso in una RSA e non può comunicare con parenti e amici. Vorrei dire una cosa al signor Carlo, che non so se può sentirmi: vede, signor Carlo,

il decreto-legge cosiddetto ristori, nel testo in esame presso questa Assemblea, prevede, con riferimento alle infrastrutture autostradali, tra cui la A22 Brennero-Modena, che le Regioni e gli enti locali interessati possano avvalersi di società *in house* nel ruolo di concessionari. Tali società hanno la possibilità di riscattare - previa delibera dell'assemblea dei soci e anche in deroga agli statuti le azioni di titolarità di soggetti diversi delle pubbliche amministrazioni. Dal momento che queste società *in house*, una volta ritornate completamente pubbliche, otterranno automaticamente il rinnovo il rinnovo delle concessioni autostradali, ritengo necessario prevedere che si occupino esclusivamente della gestione e della manutenzione delle infrastrutture autostradali esistenti e che non possano stipulare accordi di *project financing*, ovvero partecipare a società miste o ad associazioni temporanee di impresa, per la realizzazione di nuove infrastrutture. Questo per evitare che rientri dalla finestra ciò che esce dalla porta. Faccio riferimento in particolare alla società Autostrada del Brennero SpA, che diventerà completamente pubblica, ma che attualmente partecipa cento alla società ARC (Autostrada regionale cispadana), insieme all'impresa Pizzarotti & C. SpA, che ne detiene

Quest'ultima, con 37 società controllate e 42 partecipate, è fallita. È entrata in liquidazione coatta il 30 ottobre 2015, perché oberata di un passivo pari a circa 790 milioni di euro, e conta 3.700 creditori, fra cui 1.160 dipendenti o ex soci. Dei 790 milioni, 10 milioni di euro di debiti gravano sui ignari pensionati, che avevano depositato nella cooperativa parte della loro liquidazione: un buco nero da cui bisogna uscire. Signor Presidente, colleghe e colleghi, occorre che in maniera chiara l'Autostrada del Brennero SpA sia esclusa dall'Autostrada regionale cispadana. Come MoVimento 5 Stelle siamo da sempre contrari alla realizzazione dell'Autostrada cispadana, che nessun cittadino vuole, perché si tratta solo di una colata di bitume super esosa, che implicherebbe anche il pagamento di un pedaggio. La cittadinanza vuole efficienza per le strade e la viabilità ordinaria del territorio e non questi mega mostri, che servono solo ad arricchire le tasche di qualcuno e a socializzare le ingenti perdite, a spese di tutti noi cittadini. Presidente, colleghi, intervengo in quest'Aula da senatore del collegio Modena e Montagna per portarvi il grido di dolore della laboriosa comunità modenese. Nella mattina di domenica 6 dicembre si è verificata la rottura dell'argine del fiume Panaro nei pressi di Gaggio. circostanza ha costretto 360 persone a essere evacuate non solo da Castelfranco Emilia, ma anche dalla vicina Nonantola. Ad oggi, le persone sfollate sono ancora 61 e altre 300 sono rientrate a spalare il fango nelle loro abitazioni per presidiarle, ma ci vorranno dai tre ai sei mesi prima che queste abitazioni tornino agibili al cento per cento. Guarda caso, la zona di rottura dell'argine del fiume Panaro è a ridosso di quella che fu oggetto di analogo, tragico evento il 19 gennaio 2014. Non abbiamo davvero imparato nulla da tutto questo? Solo nel Comune di Nonantola oltre 1.800 edifici sono coinvolti e a Gaggio numerose aziende agricole sono devastate. I danni non sono ancora stati stimati, poiché solo in questi ultimi giorni se ne sta iniziando la conta. È inutile dire che si tratta di danni per decine e decine di milioni, che si sommano a quelli di soli sei anni fa. fa. Come dimenticarsi del Comune di Campogalliano, questa volta vittima del fiume Secchia? Qui si sono allagate addirittura aree di campagna che non lo erano mai state in precedenza. A differenza di altri Comuni, a Campogalliano non esiste nemmeno un vero e proprio argine del Secchia. Anche qui sono state evacuate una cinquantina di persone e cinque attività economiche vanno sott'acqua più volte all'anno e tutti gli anni. Dalla piena del Secchia del 2017 ve ne sono state almeno sette, ma le previsioni meteorologiche, già alcuni giorni prima, avevano previsto abbondanti piogge, che, associate allo scioglimento delle nevi, avrebbero dovuto far scattare controlli puntuali, che non sono avvenuti. La Regione Emilia-Romagna ha chiesto lo stato di calamità naturale, ma qui non dobbiamo più intervenire in emergenza, bensì in prevenzione. Ci sono 70 milioni non spesi in sei anni che avrebbero potuto portare il nostro nodo idraulico modenese a livelli di sicurezza ottimali. Perché non sono stati investiti? Sono undici anni che il comitato alluvionati non per caso è attivo, avanza proposte e idee, ma gli amministratori di sinistra si sono ben guardati dal lasciarsi coinvolgere. Qui del PD non c'è più nessuno e mi dispiace. Il Partito Democratico ci dice che non è il momento della polemica e si nasconde dietro la scusa del cambiamento climatico che provoca eventi straordinari, ma due eventi alluvionali quasi identici nel giro di soli sei anni non hanno più nulla di straordinario. La colpa dell'amministrazione di sinistra, che, invece di gestire l'emergenza, dovrebbe prevenirla, è evidente. Ormai lo sanno tutti che il nodo idraulico modenese composto dai fiumi Panaro, Secchia e Naviglio è di importanza strategica e la Regione Emilia-Romagna è quella a maggior rischio per la sua conformazione: alte montagne a sud e un grande fiume a nord. Bisogna mettere in sicurezza il nodo idraulico modenese e cambiare strategia, mettendo in campo barriere che nel tempo abbiano un ritorno di duecento I modenesi attendono un immediato cambio di strategia per il futuro. I montanari modenesi, in particolare, si attendono interventi seri per la manutenzione dei torrenti, delle briglie e dei ponti, la pulizia dei greti dei fiumi, meno burocrazia e più buon senso. Se ci si dimentica della montagna, prima la sua acqua e poi la sua terra scendono a valle e tragedie ancora più gravi possono avvenire. Signor Presidente, prevenire e non curare è il motto della Lega per fortuna, la Lega modenese si è già attivata nella raccolta di fondi e generi di necessità per questi infelici modenesi e a questi e ad altri volontari va il mio ringraziamento.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

recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*** *(Relazione